"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Signor Presidente, sarò velocissimo. Intervengo oggi perché ieri l'Aula era un po' deserta e non ho ringraziato i membri della Commissione, che nonostante alcuni alcuni problemi relativi ad un difetto di comunicazione, hanno fatto sì che l'*iter* nelle Commissioni riunite 2a e 10a fosse il più veloce possibile.

messa in evidenza la posizione di coloro che non sono vittime del bullismo, ma sono loro stessi bulli, per sottolineare l'importanza della prevenzione, ma, ancora prima, dell'educazione e della formazione, affinché i fenomeni di bullismo non si verifichino. Penso che sia uno dei punti determinanti e molto forti di questo disegno di legge, insieme ad altri. dal senatore Marti in Commissione ha espresso benissimo la posizione la senatrice Bucalo ieri durante il suo intervento, a cui mi riferisco

vorrei sottolineare con forza l'emendamento 1.102,

si sia cancellata una cosa tra le più importanti. Molto spesso i giovani non si aprono, si chiudono in se stessi, non parlano con i genitori, non parlano con le persone adulte e hanno bisogno di essere supportati da una figura importante come quella pedagogica

del ripristino della figura pedagogica in questa legge, che è il fatto fondamentale di intervento. Per questa ragione riteniamo

si dice di no a una figura che può intervenire a ridurre fortemente i danni che, se non capiti in tempo, si possono provocare nelle giovani generazioni. È davvero una cosa incomprensibile aver cancellato questo punto questo punto dalla legge approvata all'unanimità alla Camera. Signora Presidente, mi ricollego a quanto testé detto dal senatore Magni, perché in pratica abbiamo avuto un andamento anomalo in Commissione. Questo disegno di legge è il risultato di un lavoro trasversale svolto alla Camera, dove c'è stata un'ampia discussione, in particolare sulla figura professionale dell'educatore socio-pedagogico. Era stato presentato dal MoVimento 5 Stelle un emendamento che introduceva questa figura professionale, talmente apprezzata che anche il relatore di Fratelli d'Italia ha ritenuto di sottoscrivere questo emendamento, al quale si è aggiunto il correlatore della Lega,

comunque sono state superate. Questo disegno di legge è arrivato pulito (così possiamo dire) al Senato ed è stato invece sorprendentemente votato, in seno alla Commissione, un emendamento soppressivo presentato dal senatore Marti, con il quale si veniva quindi ad eliminare questa figura professionale, della quale la stessa maggioranza aveva sottolineato l'importanza alla Camera. Perfetto. Quindi chiudiamo la discussione in Commissione e il provvedimento arriva in Aula. Chiaramente cosa succede? Quando arriva in Aula la Commissione bilancio si esprime e il relatore non dice niente. All'improvviso il Governo, contraddicendosi contraddicendosi in Commissione con quanto aveva invece riferito alla Camera, esprime una contrarietà secca *ex* articolo 81 all'emendamento in questione. Io vorrei capire rispetto ad un *iter* lineare, con

conforme al relatore.

parere conforme al relatore.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula siamo chiamati a votare un provvedimento molto atteso, che tratta un tema, a mio avviso, molto sottovalutato. Sono felice che oggi assistano alla seduta proprio degli studenti perché il tema riguarda soprattutto loro. I dati più recenti portano alla luce numerosi casi di drammatico aumento tanto del bullismo quanto del cyberbullismo. Ciò ci costringe oggi a prendere atto di quanto sia marcato e pericolosamente in aumento un disagio sociale ormai evidente: rabbia e frustrazione si trasformano in vera e ingiustificata violenza. I casi di cronaca, come già altre volte ricordato in quest'Aula, ci raccontano di ragazzi che si accoltellano tra loro, che aggrediscono e feriscono docenti e personale scolastico. Non si tratta più di fastidiosi scherzi tra ragazzi. Io non posso non ricordare Io non posso non ricordare che ai tempi in cui andavo a scuola io stessa dovetti fare i conti con i bulletti del liceo. A quei tempi però i ragazzi per dispetto rubavano lo zaino...

Il tema sembra marginale, ma marginale non è. Non si tratta più di fastidiosi scherzi tra ragazzi. Voglio ricordare - lo devo anche a me stessa - che ai tempi in cui andavo a scuola, anch'io dovetti fare i conti con i bulletti del liceo. A quei tempi però si trattava di dispetti di compagni di scuola che rubavano lo zaino, strappavano i giubbotti, bucavano le ruote del motorino, deridevano qualche compagno che portava gli occhiali o spesso prendevano di mira i ragazzi con disabilità, che erano le prede più ambite. Altre volte ti deridevano non solo per giorni o per mesi, addirittura anche per anni, se ti presentavi a scuola con la scarpa sbagliata o con i vestiti non alla moda. Non si contano nemmeno i pettegolezzi poi che venivano diffusi in merito alle scritte improprie nei bagni delle scuole.

Scherzi innocenti? No, neanche così innocenti perché influiscono sulla crescita e sull'autostima proprio durante l'adolescenza che, come sappiamo, è il periodo in cui si tende ad amplificare tutto. Oggi è tutto diverso. tutto difficile da gestire per le famiglie, per i docenti e per il personale scolastico. Oggi, purtroppo, siamo davanti a fenomeni di vera violenza, che spesso sfociano anche in lesioni. Ci sono ragazzi che, per una stupida lite sui *social*, si accoltellano e purtroppo alcuni di questi casi portano addirittura anche alla morte. Non posso non ricordare in questa sede come è nata la legge sul cyberbullismo del 2017. Ricorderete tutti è nata dopo lo *shock* generale davanti al drammatico suicidio della quattordicenne Carolina Picchio di Novara che scelse tristemente di togliersi la vita gettandosi dalla finestra della sua cameretta. Una ragazza che non ha retto la vergogna e l'umiliazione di un video registrato a sua insaputa, diffuso prima nelle *chat* e poi sulla rete. Troppo pesante per lei leggere migliaia di commenti e insulti e la fragilità dell'adolescente ha preso il sopravvento. Lei aveva solo quattordici anni e un'intera vita davanti. Qualcuno ancora oggi, nonostante questi precedenti, ha il coraggio di chiamarle "ragazzate". Voglio ricordare che anche il tribunale per i minorenni di Torino, a seguito di una lettera di denuncia, scritta proprio da Carolina, poté celebrare di fatto il primo processo per cyberbullismo in Italia e stabilì che le condotte, anche virtuali, che hanno portato Carolina a togliersi la vita non possono essere derubricate a semplici ragazzate. È giusto anche ricordare e onorare la sua memoria, un'eredità preziosa per le nuove generazioni.

Si rivedono i compiti del tribunale per i minorenni, prevedendo incisivi interventi di carattere preventivo, tenendo conto in particolare della valorizzazione di percorsi educativi e rieducativi personalizzati, rivolti ai minori violenti, ma anche a sostegno di chi è vittima, guardando al contesto familiare e coinvolgendo sempre di più le famiglie, ampliando quindi il patto educativo di corresponsabilità. Mi sento di dire che forse abbiamo perso l'opportunità di allargare questo patto anche al terzo settore, che svolge sempre di più un ruolo importante sul piano educativo. Penso, ad esempio, al mondo dello sport. Da atleta paralimpica, prima ancora che da parlamentare, a me è capitato di incontrare spesso degli studenti e dei ragazzi con disabilità che sono riusciti a superare lo stato persistente di sottomissione e di bullismo anche grazie allo sport, trovando nuovi stimoli e ritrovando anche la propria autostima. Per questo motivo sono sempre stata convinta che dovremmo aiutare il mondo della scuola a usare il prezioso contributo offerto dal mondo sportivo, per i suoi valori educativi, soprattutto volti al rispetto per le regole e per gli altri. Infine, parliamo di rispetto. Si istituisce in questo provvedimento anche la Giornata del rispetto e di questo - permettetemi di dire - ci sarebbe davvero un disperato bisogno anche tra gli adulti. Questa Giornata, individuata nel 20 gennaio, è anche nel ricordo di Willy Monteiro Duarte, un ventunenne italiano di origini capoverdiane brutalmente ucciso a calci e pugni dopo essere intervenuto coraggiosamente in difesa di un suo amico e compagno di scuola, aggredito poco prima; un'altra vita spenta, un altro giovane ragazzo divenuto suo malgrado esempio di educazione e di altruismo. un'azione politica, culturale e sociale, volta al rispetto, all'educazione e soprattutto all'inclusione. Mi avvio alla conclusione, Presidente, ricordando che, per quanto ci riguarda, con uno scopo costruttivo - come è nostro solito fare - abbiamo provato anche a dare un contributo proponendo emendamenti di buon senso, che purtroppo sono stati respinti. Ne voglio citare solo qualcuno. Ad esempio, il testo lascia la facoltà alle Regioni di adottare il servizio di supporto psicologico agli studenti; noi avevamo chiesto di eliminare questa discrezionalità, prevedendo invece un obbligo giuridico e, quindi, degli interventi automatici e doverosi, non lasciati alle singole sensibilità. Avevamo chiesto di modificare il testo rivolgendoci anche a studenti maggiorenni; dobbiamo ricordare infatti che negli ultimi anni di liceo spesso ci troviamo davanti a ragazzi che hanno già compiuto i diciotto valorizzare le funzioni dei dirigenti scolastici, consentendo loro, laddove lo ritenessero opportuno, di intervenire nei casi più gravi fuori dall'orario scolastico. Infine, avevamo chiesto di disciplinare finalmente, con regole certe e soprattutto uniformi, anche l'uso del cellulare all'interno degli istituti scolastici. Presidente, concludo dicendo che tuttavia, nonostante siano state respinte e ignorate le nostre proposte, sono contenta del fatto che il Governo abbia dimostrato una disponibilità accogliendo un ordine del giorno con cui si chiede di attenzionare una nostra proposta di legge che va in questa direzione, un disegno di legge che chiede di verificare i dati anagrafici dei ragazzi che si iscrivono alle piattaforme *social*. Nonostante questo, comunque reputiamo l'impianto di questo disegno di legge un importante passo in avanti. Pertanto confermo il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi)*.

che, proprio in questi giorni, il Vaticano ha emesso un francobollo di commemorazione del sogno di Don Bosco. San Giovanni Bosco è stato uno dei più grandi educatori della storia dell'umanità, come sappiamo: a nove anni fece un sogno, che viene ricordato nel bicentenario, in cui vide Gesù Cristo che gli diceva testualmente con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità avrebbe dovuto far stare bene e crescere i giovani. Tradotto nel linguaggio moderno, vuol dire che non con divieti, ma con stimoli positivi si deve fare in modo che le giovani generazioni crescano in maniera equilibrata e sappiano rapportarsi reciprocamente. Questo provvedimento, sul quale il mio Gruppo sicuramente voterà a favore, soltanto un primo passo, perché dobbiamo essere consapevoli che c'è tanta strada da fare oltre a questa legge. Bisogna adattare una serie di comportamenti del nostro vivere quotidiano

che i giovani si abituino a stare insieme: stanno molto più volentieri isolati, con il cellulare davanti. Qui si tratta allora di dare proprio una sterzata e di cambiare la direzione in cui si evolve la nostra comunità.

a un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non all'ennesimo decreto-legge governativo di stampo punitivo o all'ingresso del

anche se ci sono certamente aspetti di criticità, che sono stati evidenziati ieri dalla mia collega di partito, senatrice Musolino. Ad all'accoglimento dei nostri emendamenti, che andavano nella direzione di implementare, per esempio, il tema dell'identità digitale

quindi che ci aspettavamo almeno l'accoglimento di questi due emendamenti, che andavano nella direzione di rafforzare il provvedimento.

assolutamente importanti e fondamentali nella politica della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo,

abbiamo bisogno di un'ulteriore riflessione anche nelle Commissioni competenti, che ringrazio, come pure il relatore. Abbiamo bisogno di questo perché è necessario fare il punto sul concetto di recupero di comunità. Oggi è una comunità sempre più fragile, divisa, dove il tema dell'odio e della violenza inizia dal linguaggio. Permettetemi di dire che anche noi dovremmo dare il buon esempio in quest'Aula parlamentare. Il linguaggio è fondamentale, soprattutto nel rapporto tra adulti e ragazzi. I numeri sono davvero allarmanti: gli ultimi dati che abbiamo di Save the Children, ma anche del Ministero dell'istruzione, ci dicono che ogni giorno ragazzi su dieci sono vittime di bullismo o di una forma di violenza e di odio su Internet e sui *social*. Ci vuole la massima attenzione e ciò significa che non basta una buona legge, se non creiamo le condizioni anche anche nelle singole comunità e nei territori per fare davvero il nuovo patto educativo. Era necessario anche qui introdurre il rapporto con il terzo settore, che è una gamba fondamentale all'interno della riforma del *welfare*, a cui noi crediamo in maniera convinta. C'è il tema della formazione e del reinserimento, perché molto spesso anche chi è bullo è stato a sua volta vittima di insulti, di violenza e di odio. Noi ci dobbiamo occupare, nelle politiche della prevenzione, di un prima, di un durante e di un dopo, perché noi crediamo nel recupero e nel reinserimento anche di quei ragazzi che hanno sbagliato. Quindi, bene, per esempio, forme di aiuto e di sostegno nel recupero, come il volontariato sociale, che è fondamentale. Lo dico con grande orgoglio, come Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: noi abbiamo presentato dei disegni di legge che sono stati anche accolti dal Ministero dello sport e dal Ministero della salute che vanno in questa direzione. Lo sport è fondamentale come strumento, come farmaco naturale per aiutare a costruire costruire luoghi di aggregazione e relazione per tenere i nostri ragazzi, soprattutto quelli sotto i quattordici anni, lontani dagli strumenti informatici e dai *social*. Crediamo che lo *sport* sia un farmaco naturale che debba essere introdotto all'interno di questo sistema di relazione e di socialità che noi vogliamo dare anche con questo disegno di legge. Così come tutte le forme creative, la musica, l'arte, la cultura, la bellezza del nostro patrimonio, che sono il nostro DNA nazionale, possono aiutare a creare un nuovo sistema relazionale e - permettetemi di dire - anche a ritrovare una parola magica, fondamentale per i nostri giovani: l'empatia. è costruire empatia. Quindi, bene la Giornata del rispetto il 20 gennaio, bene tutte le forme che possiamo utilizzare nei luoghi come la scuola. E mi permetto di fare un plauso ai nostri docenti che ogni giorno sono degli eroi *(Applausi)* che non dobbiamo lasciare da soli, perché si occupano dell'educazione dei nostri figli. E non serve più creare - purtroppo è quello che stiamo vedendo - conflittualità fra genitori e docenti; un tempo non era così, c'era un'alleanza molto forte. Noi dobbiamo ricostruire anche questo rapporto. Bene quindi che ci sia anche un referente scolastico in ogni scuola, che possa lanciare subito dei segnali di allarme, aiutare subito le famiglie a capire se c'è un disagio. Per esempio, uno dei primi disturbi che noi non dobbiamo considerare secondario è quello

Poi, guardate: tutto ciò che serve a contrastare le dipendenze noi lo dobbiamo mettere in atto nella politica della prevenzione. Serve investire in strutture, in servizi di aiuto, come lo dello psicologo, perché i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti vanno ascoltati. Bisogna ricostruire un nuovo patto generazionale. Spesso i nostri ragazzi sono da soli anche perché le famiglie,

un problema enorme per due anni. Noi di Italia Viva avevamo detto che l'unico luogo che non andava chiuso durante il Covid era la scuola, perché la scuola ha sempre creato relazioni, momenti di sostegno e di aiuto ai nostri ragazzi. Bene, mi avvio verso la conclusione. Signora Presidente, lo dico al Governo e a tutte le colleghe e i colleghi: spero che possa andare avanti un altro disegno di legge che noi abbiamo abbiamo messo a disposizione del Senato, del Parlamento e del Governo e che mi vede prima firmataria, quello di reintrodurre il medico scolastico all'interno delle scuole. È un altro presidio di sicurezza di prevenzione, per capire se ci sono dei segnali di allarme, in un'alleanza con il pediatra, con lo psicologo e con tutta una serie di figure di sostegno e di aiuto alle famiglie e alla scuola. Per tutti questi motivi chiaramente il nostro voto sarà favorevole. Finisco, signora Presidente, in trenta secondi con un appello, rivolgendomi in modo particolare al Governo. Ci sono - secondo me - degli strumenti a costo zero che possiamo mettere a disposizione delle scuole e delle famiglie. Abbiamo per fortuna tanti *testimonial* positivi, a partire dallo sport. Guardate la bellezza e i valori educativi, i valori sociali ed emozionali che sta creando il tennis in questi giorni, con una figura straordinaria, positiva e bella come quella di Sinner. Avere figure come un giovane di ventidue anni che va nelle scuole e parla nei luoghi di socialità. Ma ne abbiamo anche altri: pensiamo per esempio ad alcuni cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo e hanno parlato degli importanti problemi legati al bullismo al cyberbullismo. Ecco, anche la TV pubblica - è un appello che rivolgo ai *media* - potrebbe in questo caso aiutare moltissimo. Se ci sono dei *testimonial* positivi, mettiamoli nelle condizioni di poter parlare nella TV pubblica, di andare nelle scuole e di valorizzare il tanto di positivo che c'è nella nostra società. Altrimenti il messaggio negativo che sta passando è che abbiamo perso una generazione o che tutti i ragazzi giovani sono negativi. Non è così, perché abbiamo tantissimo da imparare dai ragazzi, ragazzi, ma serve un nuovo patto generazionale. Per tutti questi motivi, Italia Viva - Il Centro - Renew Europe voterà a favore di questo provvedimento. Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo, è complicato per me parlare del bullismo e del cyberbullismo, che fa parte - ohimè - della mia vita, più che politica professionale, di neuropsichiatra. Tanti sono i motivi - lo diceva la collega che mi ha preceduto - che ci fanno accendere l'interesse su questo argomento. Però evitiamo - non lo dico a lei, Sbrollini, che sento sempre volentierissimo, ma lo dico a me dico a me - di creare gabbie generazionali. Non ci sono solo i bambini e gli adolescenti vittime e protagonisti delle violenze mediatiche. Abbiamo soprattutto un'altra fascia, quella degli anziani, i quali spesso sono soli e hanno come unico strumento di comunicazione, per le ridotte capacità

Anche a loro dobbiamo pensare. Soprattutto, però, dobbiamo pensare che non esistono gabbie generazionali. Diciamoci la verità: gli adolescenti sembrano più vulnerabili e spesso lo sono. Pensavo a quando ero adolescente io, a quanti bullismi avrei subito. Per fortuna - lasciatemelo dire allora il cellulare non c'era, i *social media* non esistevano e quindi le poche aggressioni

Certo, dobbiamo reintrodurre vecchi strumenti per vivere la realtà: il marciapiede, i giochi di gruppo, l'oratorio,

modo, però, dobbiamo difendere i luoghi di socializzazione per anziani, che spesso viviamo come realtà residuali, ma non è così. Una bella partita a briscola insieme ai coetanei, magari anche a dei giovani e delle giovani, per esempio con la collaborazione del terzo settore, può essere un grande deterrente contro

veri o finti, perché nella virtualità dei *social media* è tutto vero, anche le finzioni peggiori. E questo, forse, è il danno più grave che i *social media* arrecano. È È la solitudine che genera mostri, la solitudine dei bambini, degli adolescenti, degli anziani. Come possiamo fare

per chi gestisce, spesso anche un po' irresponsabilmente, i grandi *social*. Ma non è solo questo: magari fosse solo questo. Posso fare un esempio un po' banale? Il coltello serve per affettare meravigliosi salami emiliani, ma serve anche per uccidere. Che facciamo? Eliminiamo i coltelli? No, cerchiamo di evitare le circostanze per cui un coltello è causa non di delizia, ma di delitto:

diciamoci la verità. Quando penso alla verità mi preoccupo, perché spesso la cosiddetta verità ha creato mostri, delitti e la giustificazione dei *gulag* o delle delle camere che asfissiano le persone, perché un po' diverse per una verità che non esiste. Cerchiamo una realtà compatibile con la ragione. Il vero protagonista di questi "crimini di pace", una definizione molto legata al mio 1968, di età ma anche in parte di appartenenza, è il popolo dei silenziosi, il popolo di chi non reagisce, il popolo di chi è complice, nel proprio silenzio, di questi crimini di pace. Diciamoci la verità: la persona che violenta una persona fragile lo fa perché, accanto alla sua proposta indegna di comunicazione mediatica, cento, mille, centomila o un milione di altre persone accendono la loro attenzione e danno forza a chi delinque senza dare nulla di positivo, senza dire "hai sbagliato"; anzi, con il silenzio partecipante diventano i complici peggiori. Certo, signor Presidente, dobbiamo dire sì, anche con serenità, ma con gioia no, perché quando c'è un delitto non siamo mai gioiosi; ci sentiamo sempre un po' complici, con i nostri silenzi, con la voglia di fare perché non riusciamo a fare. Ma anche in quest'Aula: io, con il problema di dove mi devo mettere con il mio il mio *scooter*, qualche volta credo di bullizzare occupando spazi impropri; anzi, sarà un argomento che riproporrò. Credo che sia il silenzio che uccide.

a qualunque età appartengano. Soprattutto, dobbiamo agire in maniera dolce, ma fortemente educativa, perché si rompa il clima del silenzio, la complicità deleteria che viviamo in questi giorni. Non è periodo di progressi, non è periodo di colpevolizzazione; è il periodo del coinvolgimento attivo. Questo propone la legge e non può non vederci complici positivamente di dare un voto positivo. Un ultimo punto: si parla del tribunale dei minori e di maggiore attenzione alla voce dei bambini. Lancio un appello: costruiamo un percorso per istituire il tribunale delle famiglie *(Applausi)*, dove davvero si dia spazio a tutte le voci di questa complessa realtà che rimane, però, unico punto di riferimento concreto della nostra realtà. Grazie e viva la vita.

un uso improprio della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti. I ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei diversi per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o l'essere stranieri. Il bullismo è associato a problemi di salute nel periodo adolescenziale:

La cronaca ci dà conto, quotidianamente, della pervasività del fenomeno e della sua pericolosità. Dietro ogni atto di violenza - il bullismo è violenza - ci sono ragazze e ragazzi che soffrono. Gli studi riferiscono che all'interno delle famiglie con il crescere dell'età diminuisce la facilità di avere un rapporto coi ragazzi, che difficilmente si aprono con i propri genitori. Così è usuale che la vittima del bullismo e del cyberbullismo abbia difficoltà a parlarne in famiglia, a raccontare ciò che vive. Tant'è che esiste un'enormità di casi sommersi e si ha più difficoltà a contrastare il fenomeno. Proprio in ragione delle difficoltà dei ragazzi a confidarsi con i propri genitori, è importante intervenire nel contesto scolastico, che rappresenta l'ambiente naturale, il luogo in cui si svolge la maggior parte della vita sociale degli adolescenti. A questo proposito occorre tener presente che numerosi studi indicano anche un'associazione fra l'essere stato vittima di bullismo e l'abbandono scolastico. Ovviamente i testimoni testimoni (genitori, insegnanti, amici) sono figure che hanno un ruolo potenzialmente decisivo per intercettare, sostenere e interrompere un'azione fisicamente e psicologicamente dolorosa. Per tale ragione è necessario realizzare azioni realizzare azioni di prevenzione e di intervento precoce, utilizzando la scuola come contenitore privilegiato di tale azione. È dimostrato, infatti, che i trattamenti più efficaci per le condotte antisociali riguardano lo sviluppo di competenze emotive e relazionali attraverso attività scolastiche che iniziano precocemente, fin dall'età infantile e preadolescenziale. Ciò consente di prevenire fenomeni di discriminazione, marginalità sociale e persecuzione in ambito scolastico, che possono dar luogo a forme di aggressività e incidere irrimediabilmente sulla personalità e sulla salute mentale delle vittime. Fatta questa premessa, dico subito

intervenire subito su un problema che riguarda tantissime persone, per lo più giovanissimi e giovanissime. Soprattutto spiace che siano stati approvati in Commissione emendamenti che ne hanno depotenziato la portata innovativa. L'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo deve infatti essere prioritariamente di natura educativa e pedagogica. L'emendamento 1.3, a firma del senatore Marti, approvato in Commissione sopprime invece all'articolo 4-*bis* il servizio di sostegno psicologico agli studenti e il servizio di coordinamento pedagogico, amputando così in maniera incomprensibile l'intento originario del disegno di legge basato non sulle azioni repressive,

la scuola svolge un ruolo importante. Se i ragazzi hanno difficoltà ad aprirsi con i propri genitori e i propri familiari, è necessario avere una figura che non può che essere psicologica e pedagogica dentro la scuola.

sono motivate da tali ragioni. Ad ogni modo il giudizio sul testo di legge che abbiamo dato è positivo e speriamo che giunga velocemente all'approvazione. Pensiamo che questo disegno di legge sia un primo passo ed è per questa ragione che il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà

il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare rappresenta un passo cruciale nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Oggi diamo un segnale di unità del Parlamento, un segnale che rappresenta il miglior messaggio per dimostrare quanto le istituzioni siano attente e decise a fornire gli strumenti più efficaci per combattere e sconfiggere un fenomeno drammatico e sempre più dilagante. Parliamo di un flagello che minaccia quotidianamente l'integrità, il benessere emotivo e, troppo spesso, anche la vita stessa dei nostri giovani. Questi fenomeni sono veri e propri attacchi alla dignità individuale, lasciano cicatrici e, a volte, danni irreparabili nella mente, nel cuore e nell'anima dei bambini e degli adolescenti. Parliamo di una piaga sociale, di un *virus* subdolo che continua a mietere vittime, soprattutto fra i più giovani. Il bullismo - come sappiamo - è sempre esistito. Quelli della mia età se lo ricordano già descritto nel libro «Cuore». Chi non ricorda Franti, il bulletto senza rispetto per niente e per nessuno? Quando però non esisteva la rete, quella vessazione continua, quell'umiliazione, quella sensazione di pericolo cessava appena si cambiava ambiente, tra le braccia dei familiari, protetti dalle mura domestiche. Oggi non è più così: viviamo in un'epoca dove una parola o un'immagine possono diventare armi micidiali perché veicolate proprio con la rete. Crollano le barriere di protezione. Basta accendere il telefonino ed essere connessi per non trovare più pace da nessuna parte. Le vittime vengono raggiunte in ogni singolo momento della loro giornata e in ogni angolo, in ogni rifugio, anche quello della propria casa. Il provvedimento di oggi rappresenta anche una bussola necessaria per navigare nelle acque agitate di una società digitale, in cui il cyberbullismo si manifesta con una virulenza e una pervasività senza precedenti. Con questa legge interveniamo e lo facciamo in continuità con il lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ho avuto l'onore di presiedere. Ricordo il *dossier* che riassume 3 P: prevenzione, protezione e punizione. Sappiamo che questi fenomeni si combattono con la forza gentile, più sottile ed efficace della prevenzione, con l'educazione e la cultura dei valori e del supporto. La punizione interviene infatti quando c'è già una vittima, c'è già sofferenza e quando magari è già troppo tardi. La famiglia deve tornare ad avere un ruolo primario, quale primaria agenzia educativa e non solo per l'articolo 30 della Costituzione, che riconosce il diritto e dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, ma perché è tra le mura domestiche che si cominciano a formare i nostri figli, che magari si cominciano a intravedere segnali di disagio o comportamenti aggressivi. La famiglia deve essere il primo e il più influente contesto educativo nel quale vengono trasmessi valori come il rispetto, l'empatia, la responsabilità e l'esempio personale. incoraggiare una comunicazione aperta, onesta e vitale, così come è vitale parlare regolarmente di ciò che accade a scuola e *online*, perché aiuta i genitori a rilevare eventuali segni. importante è monitorare l'uso dei dispositivi digitali, essere consapevoli dei siti che frequentano, delle app che utilizzano, degli amici con cui interagiscono. Insegnare ai bambini come navigare in sicurezza, compresa la gestione della *privacy*, il riconoscimento delle potenziali truffe e le strategie per affrontare il cyberbullismo, è fondamentale. Ma in troppi casi si verifica una dolorosa verità: genitori che, di fronte ai segnali allarmanti dei comportamenti dei propri figli, scelgono di non vedere, di non accettare o di minimizzare la gravità delle azioni del proprio bambino. «Non può essere mio figlio», «dai, è solo un gioco tra ragazzi»: sono frasi che abbiamo sentito spesso, espressioni di un rifiuto che contribuisce alla perpetuazione del ciclo di sofferenza. Questo atteggiamento di negazione non solo impedisce un intervento precoce, ma contribuisce anche a un senso di impunità, che alimenta la ripetizione nei confronti degli altri, delle vittime. Minimizzare il problema da parte dei genitori trasmette un altro messaggio pericoloso: che le azioni commesse non hanno conseguenze serie e che non è necessario rispettare l'altro. Il nostro disegno di legge si propone di intervenire anche su questo fronte, proponendo campagne di sensibilizzazione rivolte esplicitamente ai genitori, affinché possano riconoscere i segni di un comportamento problematico. Verranno forniti gli strumenti pratici su come agire in queste situazioni, incentivando un approccio costruttivo, che vede i genitori non come giudici severi ma come guide responsabili nel processo di crescita dei loro figli. Subito dopo la famiglia tocca ad un altro presidio fondamentale, la scuola, le scuole; è al loro interno che si verificano più frequentemente gli atti di bullismo. Il loro ruolo è strategico per fronteggiare questa piaga, perché hanno gli strumenti per l'emersione, il monitoraggio, la segnalazione. La scuola deve essere un luogo di ascolto attivo, pronto a intervenire, non con l'accusa ma con il supporto. Il provvedimento introduce il concetto di responsabilità condivisa, riconoscendo il valore e il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica nel suo complesso, inclusi gli studenti, gli insegnanti e anche i dirigenti. È fondamentale la figura del docente referente, che agirà come ponte tra la scuola e la famiglia. La formazione specifica del personale scolastico mira a creare una prima linea di difesa. L'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio all'interno delle scuole, che vede la partecipazione di studenti, insegnanti ed esperti, è sicuramente un passo innovativo verso la costruzione di un ambiente educativo in cui ciascuno si senta responsabile del benessere degli altri. Inoltre, le direttive per le scuole verranno aggiornate ogni due anni, misura vitale per rimanere al passo con l'evoluzione di un fenomeno in rapida trasformazione. Il cyberbullismo, poi, impone una più ampia riflessione sui problemi connessi all'uso della Rete. Bisogna contrastare l'uso anonimo della rete Internet. Molti utenti si nascondono dietro l'anonimato della rete attraverso profili falsi e hanno condotte aggressive che magari nella vita reale non avrebbero, per vergogna. È necessario quindi il coinvolgimento degli operatori di rete, promuovendo la creazione di un vero e proprio codice di etica digitale. Tuttavia, mentre tracciamo questi percorsi di prevenzione, dobbiamo affrontare la dolorosa realtà che alcune ferite sono state già inferte. Per le vittime il nostro disegno di legge prevede un supporto psicologico, un faro di speranza per guidarle fuori dalle tenebre del trauma. Solo attraverso l'accompagnamento potremo sperare di mitigare i disagi e le sofferenze causate alle vittime, alle vittime, offrendo ai giovani gli strumenti per superare le difficoltà e rafforzare anche il loro percorso di crescita. In questa tragedia, purtroppo, le vittime sono tutti gli attori: chi perché lo subisce, chi perché vessato, chi perché non ha avuto la fortuna di poter contare su un contesto familiare sano, attento, protetto, non violento, perché vive in un contesto di disagio. Vittime, sì; anche loro vittime di una mancanza di di cultura, spesso costrette a vivere dove vige la legge del più forte, senza che possano contare su strumenti o famiglie solide. Mi avvio alla conclusione: non possiamo etichettare i bulli come persi dalla società; anche loro necessitano di un cammino di rieducazione per comprendere la gravità dei loro atti e apprendere il rispetto per l'altro. Per questo la legge prevede percorsi educativi e riabilitativi, monitorati dai servizi sociali. Con il voto di oggi dimostriamo che non ci si può limitare alle sole parole di circostanza in occasione di una ricorrenza, ma rispondiamo con i fatti al grido d'aiuto di tanti, troppi giovani, che spesso si sentono soli nell'affrontare una battaglia più grande di loro. Noi ci schieriamo al loro fianco, tendiamo loro una mano e li accogliamo tra le braccia sicure di uno Stato chiamato a fare ogni sforzo possibile per proteggere i più deboli. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

sicuramente penserei a quella di Penelope, la moglie di Ulisse. Il perché è presto detto: nella seduta del 28 giugno 2023 delle Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera, durante l'esame del disegno di legge che oggi è oggetto dei lavori di quest'Assemblea,

e ulteriormente sottoscritta da una collega di Fratelli d'Italia. Successivamente è intervenuta anche la correlatrice, una deputata della Lega, dichiarandosi convintamente a favore della riformulazione proposta. Dopo l'espressione del parere favorevole anche del Governo, nella persona del vice ministro Sisto, si è aperto un breve spazio di discussione, nel quale la collega D'orso si dichiarava molto soddisfatta della riformulazione, poiché coglieva appieno - per una volta, aggiungerei - lo spirito dell'emendamento da lei proposto. Interveniva poi in dichiarazione di voto l'esponente di "Fratelli del Nord Italia" che aveva sottoscritto l'emendamento, manifestando entusiasmo per la certa approvazione del testo, poiché - cito testualmente

Anche Forza Italia annunciava il proprio voto favorevole e, una volta posto ai voti, l'emendamento è stato approvato. Veniamo a noi:

Voi, come maggioranza e Governo, non sapete cosa fa la mano destra rispetto alla sinistra. Ritornando all'Odissea, rappresentate proprio il mito di Penelope,

e di notte disfate. Siete l'incoerenza fatta maggioranza e state legiferando in maniera schizofrenica sulla giustizia.

abbandonando il profilo penalistico, già inizialmente residuale, per privilegiare un approccio prevalentemente educativo e preventivo e lasciare ad altre sedi gli interventi di carattere repressivo (e questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo). I numeri relativi a chi ha subìto o assistito a episodi di bullismo e cyberbullismo sono in costante aumento e il mondo degli adulti non può più ignorare questa realtà, minimizzandola o normalizzandola. Questa proposta, frutto dell'ascolto di magistrati, di avvocati minorili, di dirigenti scolastici, di servizi sociali minorili, di docenti ed educatori, mira a coordinare tali sforzi, superando una concezione di interventi settoriali. La creazione di una rete efficace è il concetto chiave di questa legge, con l'obiettivo di bilanciare prevenzione e contrasto in modo armonico. Si è esteso il perimetro di intervento della già legge n. 71 del 2017, che di certo ha avuto il merito di portare all'attenzione di questo Parlamento e della società tutta il problema del cyberbullismo, introducendo il fenomeno del bullismo, dando finalmente anche una definizione di cosa sia il bullismo, perché se è vero che i due fenomeni non sono del tutto sovrapponibili e hanno alcune caratteristiche, appunto, differenti, è pur vero che la dinamica relazionale che si instaura è identica. Vi è da una parte un prevaricatore e dall'altra una vittima, che viene umiliata ed emarginata dal contesto dei pari attraverso atti di violenza fisica, verbale e psicologica. Dunque, è possibile, anzi è opportuno affrontare con una strategia unitaria i due fenomeni che spesso vanno a braccetto. Con questa proposta, quindi, rafforziamo il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ampliando il novero dei soggetti qualificati chiamati a farne parte e prevedendo che venga convocato con cadenza semestrale. Prevediamo che le linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, adottate dal Ministero dell'istruzione, indichino vere e proprie procedure operative di cui ogni istituto dovrà dotarsi, recependole nel proprio regolamento interno. In pratica, vi dovranno essere protocolli di base uniformi per tutte le scuole, da attivare nel momento in cui è segnalato o emerga un episodio di bullismo o cyberbullismo, o una situazione di dipendenza, in modo che non gravi sul dirigente scolastico, da solo, la scelta su come agire; una scelta che diviene altrimenti, oltre che assai gravosa sotto il profilo umano, anche assai discrezionale e diversificata da scuola a scuola, mentre riteniamo che la risposta degli adulti debba essere sempre coerente, prevedibile ed equa per essere compresa, oltre che autorevole. Il cuore di questo disegno di legge è che intendiamo intensificare la sinergia tra scuola e famiglie e a questa finalità rispondono anche altre disposizioni, come quella di inserire nel cosiddetto patto di corresponsabilità l'impegno da parte delle famiglie a partecipare attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete Internet e delle comunità virtuali, affinché sappiano quanti rischi oggi riservano ai nostri giovani e collaborare - sottolineo collaborare - con la scuola per l'emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, ma anche delle situazioni di uso e abuso di alcol, di sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza, tra cui oggi possiamo annoverare anche la nomofobia. Poi, ancora, non ci siamo sottratti alla necessità di fornire una risposta forte ed efficace innanzi alle condotte più gravi e reiterate di bullismo, ma anche dinanzi a tutte le forme di devianza minorile, adattando al contesto attuale le cosiddette misure rieducative del tribunale per i minorenni ed introducendo i percorsi di mediazione che hanno l'obiettivo di ricucire la relazione tra il bullo e la vittima. Quando mancano le condizioni per attivare la mediazione, perché, ad esempio, la vittima non presta il consenso, il tribunale, solo in quel caso, potrà disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative, sotto la direzione dei servizi sociali. Tutti questi progetti dovranno essere come abiti tagliati su misura per il ragazzo o la ragazza che ne siano destinatari e dovranno avvalersi di certo delle associazioni di volontariato e del terzo settore, perché spesso fare un'esperienza nel volontariato o comunque nel sociale può essere più formativo e performante di tante altre iniziative. Con un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera è stato esplicitato anche il progetto di intervento educativo che potrà prevedere la frequenza - l'abbiamo sottolineato prima e c'è stato creativa, di musica o di attività sportive, insomma tutte quelle attività capaci di canalizzare l'aggressività, di insegnare come fare squadra e di sviluppare percorsi di introspezione capaci di offrire opportunità a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari, per il contesto di provenienza, hanno poche opportunità di crescita culturale e ancor meno possibilità e occasioni di scoprire un proprio talento. Presidente, mi avvio alle conclusioni. Perché vi dico questo? Perché a volte, per recuperare un disagio e per strappare un adolescente a dinamiche relazionali malsane o a una dipendenza può essere sufficiente far intravedere che esiste un'alternativa migliore, può essere sufficiente far comprendere che si può essere persone migliori. L'auspicio è proprio che la cassetta degli attrezzi che questo provvedimento intende fornire possa servire ad evitare a quanti più giovani possibile le ferite che del bullismo, sia agito, sia agito, sia anche subito, i cui effetti si portano per tutta la vita. Per tutte queste ragioni, nonostante qualche incidente di percorso in Commissione, esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Grazie Presidente, grazie colleghi. Purtroppo i fenomeni che stanno coinvolgendo i nostri ragazzi destano veramente grande preoccupazione. Non occorrono delle volte i numeri; però, se guardiamo il monitoraggio che è stato fatto dal Ministero dell'istruzione, è emerso che sono aumentati i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, uno del 22 e uno del 27 per cento rispetto agli anni precedenti. Se guardiamo anche a un sondaggio, risulta praticamente che il 27 per cento dei ragazzi dichiara di aver subito atti di bullismo e il problema è che il 17,5 per cento dichiara di aver commesso atti di bullismo. Sono numeri che si accostano e che preoccupano. Le motivazioni per le quali ci troviamo di fronte a una gioventù così in difficoltà in difficoltà probabilmente non le riusciremo a sviscerare, di certo non oggi, forse neanche in questi tempi; forse qualche studio permetterà di individuare la causa per riuscire ad estirpare questa mala pianta. Di certo il disorientamento anche una crisi sociale che ha coinvolto veramente la famiglia e il futuro o forse anche un momento di transizione verso un qualcosa che non sappiamo e che non conosciamo. Teniamo anche presente una grossa problematica che riguarda la prima generazione di stranieri stabiliti che a volte in cerca della loro identità. Questo disegno di legge si innesta su un percorso che è già stato inaugurato da questo Governo, volto ad affrontare i temi dei ragazzi, ma anche quelli delle devianze più estreme sulla delinquenza minorile, come è stato fatto con il decreto Caivano, che ancora ricordiamo. Non cesseremo mai di sottolineare la bontà di quel provvedimento, il quale ha previsto delle norme e delle innovazioni sul processo minorile, ma ha anche percorsi di reinserimento e di rieducazione civica e sociale del minore. inoltre sdoganato degli istituti che sono al di fuori del processo: l'avviso orale, l'ammonimento, il divieto di utilizzare alcuni strumenti (i telefoni) nel caso in cui si incorra in alcuni episodi. Ma non si parla solo di delinquenza; stiamo parlando qui di bullismo e di cyberbullismo. Non possiamo nasconderci dietro a un dito, perché a volte i fenomeni di bullismo non sono che un preludio, poi, a percorsi più gravi e a condotte magari più

Questo disegno di legge estende il perimetro dell'applicazione della legge del 2017 sul cyberbullismo, andando a prevedere figure e percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo in tutte le sue manifestazioni, così agendo con delle strategie di attenzione e tutela dei minori, che devono essere visti non solo come vittime, ma anche come responsabili di illeciti.

un piano di azione integrato con tavoli tecnici, prevedendo anche delle sinergie. Qui è importante che vi siano sinergia e coordinamento fra i servizi socio educativi, il territorio, le scuole, gli enti locali, gli enti sportivi e gli enti del terzo settore. Dobbiamo veramente consolidare la nostra comunità attorno a questi ragazzi e creare per loro l'ambiente per poter crescere sani e in serenità.

di monitoraggio, dove, anche qui, vengono inseriti i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti, per creare un coordinamento, per riuscire a non solo a fare dei monitoraggi, ma ad elaborare anche delle strategie. Per quanto riguarda il mondo della scuola è stato molto interessante l'accoglimento dell'emendamento del presidente Marti, che veramente ringraziamo, il quale è proprio volto a eliminare una problematica che poteva creare una sovrapposizione di competenze fra il servizio di coordinamento pedagogico e la previsione del servizio psicologico. Quello cui noi dobbiamo guardare, colleghi, non sono le burocrazie, non è la creazione di istituti, enti e tavoli, ma la creazione di un sistema efficiente, che vada ad incidere sulle attività svolte e che non vada, invece, a frenare o bloccare alcuni percorsi virtuosi. Quindi, veramente un

è la prima comunità, dopo la famiglia, ad accogliere il cittadino che sta crescendo e quindi ha una grandissima capacità di formarlo. Importantissimi, poi, sono stati altri interventi,

quanto introdotto in questo provvedimento, che va a prevedere anche degli strumenti straordinari, quali il percorso di mediazione oppure l'adozione di alcuni progetti educativi, portando i ragazzi a partecipare a laboratori teatrali, di scrittura, di musica, di attività sportiva, artistica: artistica: quelle attività che veramente sono idonee a far maturare anche un sentimento di rispetto nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di se stessi. Quindi, non possiamo che concludere sottolineando ancora il forte convincimento della Lega a supportare e dare il proprio voto positivo nei confronti di questo provvedimento, ricordando e anche sottolineando la bontà delle iniziative e delle attività che sta portando avanti il ministro dell'istruzione Valditara, che sta veramente delineando un ruolo diverso e importante

il dibattito su questo disegno di legge rappresenta davvero un momento molto importante, perché offre a tutti noi l'occasione di essere protagonisti per approvare una legge giusta a difesa dei più giovani. Il bullismo e il cyberbullismo sono un uragano di violenza un uragano di violenza e sopraffazione che entra nella vita delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e crea gravissimi danni alla loro crescita. Prima era solo il bullismo, poi con la veloce diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie (il *web* e gli *smartphone)* questi fenomeni hanno assunto una nuova forma dentro quel fenomeno che oggi chiamiamo cyberbullismo. Perché serve questa legge? Perché il fenomeno del bullismo rappresenta, come dicevo già prima, una grave forma di violenza che interessa in particolar modo i giovani. Nel caso del cyberbullismo sono i *social* che rappresentano il principale canale in cui si fanno strada le violenze, seguiti da *chat*, messaggi e videogiochi *online*. c'è un fatto che in questa discussione non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento del numero dei casi di cyberbullismo, in particolare. Anche in questo caso abbiamo moltissime statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento. La maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile, con conseguenze psicofisiche che vanno dal mal di testa ai dolori allo stomaco e che si manifestano con mancanza di appetito o disturbi del sonno. Questi fenomeni, che risultano essere molto diffusi nei Paesi ad alto reddito, richiedono un intervento politico politico efficace e misurato, proprio perché la loro diffusione provoca effetti dannosi sull'apprendimento e sul comportamento dei minorenni, tali da ridurre l'efficacia degli investimenti pubblici nell'istruzione e nel benessere dei bambini di ogni Paese. C'è C'è un dato che deve essere considerato, a mio parere: secondo uno studio dell'Istituto degli innocenti, infatti, solo il 5 per cento delle vittime di cyberbullismo lo segnala alle autorità competenti. Allora come si contrasta questo fenomeno? Si contrasta - forse va detto proprio in modo chiaro - attraverso una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione, famiglie, scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, associazioni sportive, Forze dell'ordine, tribunali dei minori. Soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Noi - lo voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato - in questa discussione stiamo facendo la nostra parte, per la prima volta cercando una condivisione che, su un tema sensibile come il bullismo e cyberbullismo, diventa un imperativo etico e non solo politico. Abbiamo bisogno di completare il quadro normativo dopo l'entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, anche perché pensiamo che il bullismo e il cyberbullismo siano fenomeni strettamente legati tra di loro, e sarebbe stato un errore disciplinare in due contesti normativi differenti due fenomeni che invece sono strettamente connessi tra loro. Signor Presidente, mi lasci ricordare in quest'Aula il grande lavoro svolto dalla senatrice del PD Elena Ferrara nella XVII legislatura. È grazie a lei se siete arrivati nel 2017 ad approvare approvare una legge contro i fenomeni di bullismo. Si aggiunga anche che la legge n. 71 del 2017, proprio grazie a quel lavoro, è stata largamente condivisa tra le forze politiche e i soggetti istituzionali del mondo scolastico ed educativo, dunque sarebbe stato un errore non averla come riferimento oggi. Quella legge, fortemente voluta dal Partito Democratico, ha avuto il merito di introdurre misure specifiche di contrasto al fenomeno, che oggi possono essere integrate dal dispositivo di cui stiamo dibattendo, maggiormente orientato sul ruolo della prevenzione e delle famiglie. Signora Presidente, non mancherà il nostro sostegno a questo disegno di legge, lo dico con chiarezza, ma certo siamo rimasti delusi dal comportamento adottato da questa maggioranza. In Commissione sono emerse le ambiguità e le scorrettezze di chi prima ha lasciato credere di voler andare celermente in Aula e poi ha consentito l'approvazione di un emendamento della maggioranza che posticipa ancora i tempi per approvare il disegno di legge, rinviandolo a una terza lettura. Vi siete accorti con un certo ritardo che nell'*iter* parlamentare non sono state inserite le necessarie coperture e non lo avete nemmeno detto. Si sarebbe dovuto intervenire subito, evitando di allungare i tempi e mancare un obiettivo che avrebbe dato ancora più senso alla nostra azione, cioè approvare questa legge nella giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, che abbiamo celebrato anche in quest'Aula lo scorso 7 febbraio. La cosa ancor più grave è che si è pensato di trovare le coperture che non c'erano, cancellando la figura del coordinatore pedagogico, i cui frutti sono davanti a tutti, come abbiamo visto. È una figura importante che ha agito bene nelle scuole in questi anni. Ho sentito le giustificazioni che ha dato ieri nel suo discorso la senatrice Bucalo, ma la verità è che le coperture mancanti, che hanno costretto la maggioranza ad andare in terza lettura, si sono trovate attraverso la cancellazione di questa figura

Tra gli elementi di forza del disegno di legge in esame, che nasce anche da una proposta del Partito Democratico, c'è la creazione di un sistema di segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo, che consenta agli studenti di denunciare i comportamenti aggressivi, subiti o osservati. Questo sistema potrà essere gestito da figure specializzate all'interno delle scuole, che si occuperanno di verificare la veridicità delle segnalazioni e di adottare le misure necessarie per contrastare il fenomeno, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Per quanto riguarda le misure rieducative, il disegno di legge prevede l'istituzione di un servizio di assistenza e supporto psicologico per i minori coinvolti in comportamenti aggressivi, al fine di favorirne la rieducazione e il reinserimento nella società. Si prevede inoltre la possibilità di adottare misure alternative alla detenzione per i minori autori di reati di bullismo, con il sostegno dei servizi sociali territoriali e il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tra le modifiche spicca soprattutto l'intervento legislativo in materia penale. La modifica, attesa da tempo, prevede all'articolo 1 l'intervento sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo

Già attualmente la giurisprudenza, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare negli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Con questa proposta normativa sarà sarà però finalmente disponibile un chiaro ed esplicito quadro normativo, visto che le stesse sanzioni previste dalla legge n. 71 del 2017 per il cyberbullismo vengono estese, all'articolo 1 del testo in discussione, anche ai casi di bullismo. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione ricordando che nel 2023 è stata presentata una ricerca interessante di Telefono azzurro, condotta in collaborazione con Doxa Kids. uno studio su adulti e adolescenti nel mondo digitale che descrive in maniera drammatica il profondo cambiamento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali. Il bullismo rappresenta uno dei fenomeni più temuti dagli adolescenti e, tra le preoccupazioni maggiori, c'è proprio la condivisione pubblica di dati personali, minacce, timori, paura di condividere luoghi e momenti. Il bullismo e il cyberbullismo sono una grave minaccia ad uno sviluppo sereno dei minori e degli adolescenti. È per questo che ritengo che le novità introdotte da questa proposta di legge rappresentino un passo in avanti concreto che noi, tutti insieme, dobbiamo compiere per assicurare un futuro più giusto alle giovani e ai giovani del nostro Paese. È per queste ragioni e per il fatto che si è visto un approccio diverso della maggioranza rispetto a quello avuto nel passato, ad esempio, sul decreto Caivano, che annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

colleghi, i bambini non sono intelligenza artificiale, bisogna ascoltarli, accompagnarli e difenderli. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda la vita di migliaia di bambini violati e, nei casi più gravi, uccisi da un nemico invisibile o difficilmente individuabile perché si nasconde dietro un alleato fortissimo che è la rete. Questo provvedimento ci rende orgogliosi non solo perché è una misura che ha trovato un consenso trasversale, perché tutela i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti e le famiglie, facendo sentire la presenza dello Stato affinché le vittime non siano più sole. Oggi è quindi sicuramente una giornata importantissima. La proposta finale del provvedimento, sintesi di diverse proposte di Fratelli d'Italia e delle altre forze politiche, dota il nostro ordinamento di una legislazione in materia di contrasto del bullismo e del cyberbullismo probabilmente tra le più efficaci e complete in Europa. Considerata la dimensione sempre più ampia di questo fenomeno, che va di pari passo all'utilizzo smisurato e poco controllato, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi dei *social*, serviva costruire una legge che applicasse una serie di misure per la prevenzione, la rieducazione e che coinvolgesse tutta la comunità educante. Proprio partendo dalla legge n. 71 del 2017, in materia di di cyberbullismo, abbiamo apportato delle misure di prevenzione del fenomeno, codificando la materia con una definizione chiara. chiara. Abbiamo dotato infatti ogni istituto scolastico di un codice interno di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo *(Applausi)*, permanente di monitoraggio e di strumenti adeguati di sostegno psicologico agli studenti, con l'intento di coinvolgere il minore in un progetto educativo che può concludersi con un esito positivo e, in mancanza di questo, prevedere l'affidamento del minore ai servizi sociali e, nei casi ancora più gravi ed estremi, il collocamento del minore in una comunità. Sono misure preventive che, esulando dall'ambito strettamente penale, possono consentire anche una applicabilità ai ragazzi *under* quattordici, al di fuori cioè della soglia di imputabilità. Inoltre, abbiamo previsto una delega al Governo entro dodici mesi per emanare i decreti attuativi su alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio l'attivazione dei servizi di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche, piattaforme di formazione e di monitoraggio e un potenziamento del servizio per l'assistenza alle vittime, anche con il numero pubblico e gratuito, il 114, che potrà essere utilizzato per chiedere aiuto in tempo reale. Abbiamo introdotto un'altra importante misura, quella della responsabilizzazione dei genitori per i danni cagionati dai figli minori nell'utilizzo delle piattaforme informatiche e telefoniche, intervenendo sui contratti dei fornitori. In aggiunta a questo, ci saranno importanti campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione. quindi introdotto una serie di misure significative di prevenzione, di emersione del fenomeno, di sensibilizzazione e di educazione, oltre che di assistenza e supporto psicologico.

dicendo che esiste già nella scuola: è in capo ai dirigenti scolastici, che si avvalgono della collaborazione dei docenti referenti. *(Applausi)*. come al solito, anche quando c'è una condivisione, di una polemica inutile e inappropriata. Concludo. Quando si ha a che fare con materie così delicate anche una buona legge come questa non basta se non vi è un cambio di passo culturale e sociale. Questa proposta è un tassello che si colloca proprio in questa ottica. ottica. In conclusione, esprimo convintamente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole, rivolgendomi ai tanti ragazzi, alle famiglie e alle persone più fragili vittime di bullismo, di

e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ricordato dall'onorevole interrogante, nell'ambito della riprogrammazione del PNRR, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha chiesto e ottenuto risorse per due miliardi di euro per la nuova misura PNRR, che istituisce un fondo rotativo per i contratti di filiera. Ricordo che la misura dei contratti di filiera trova la sua attuale fonte finanziaria nel Piano nazionale per gli investimenti 1,203 miliardi di euro, ripartite su diverse linee di intervento, e in particolare 690 milioni di euro per il quinto bando (contratti di filiera settore agroalimentare), 350 milioni di euro per lo scorrimento del quarto bando (contratti di filiera settore agroalimentare), 103 milioni di euro per i distretti del cibo, 50 milioni di euro per il primo bando (contratti di filiera settore pesca e acquacoltura), 10 milioni di euro per il primo bando (settore forestale). Lo strumento finanziario introdotto con il PNRR è innovativo rispetto al passato e prevede la concessione di contributi sia nella forma del fondo perduto

un'apposita convenzione tra l'Ismea e il MASAF, che recherà anche la disciplina delle modalità di gestione del nuovo Fondo. Le risorse aggiuntive, pari a due miliardi di euro, saranno successivamente destinate allo scorrimento delle graduatorie esistenti per il quinto bando e per il primo bando (contratti di filiera settore pesca e acquacoltura e settore forestale). Si tratta di tre misure verso le quali le imprese del settore agricolo hanno dimostrato un grande interesse. Infatti, per il quinto bando (contratti di filiera agroalimentare) la graduatoria definitiva di cui al decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023 ha registrato un *overbooking* di oltre quattro miliardi di euro. Analogamente, il bando per i contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura ha registrato, per i soli contratti che non necessitano di notifica e di aiuto individuale e di cui alla graduatoria del decreto n. 399082 del 28 luglio 2023, un *overbooking* di oltre 30 milioni di euro. A questi si aggiunge, ai progetti per i quali è necessaria la notifica individuale, un'ulteriore *overbooking* di quasi 40 milioni di euro. Anche il bando relativo ai contratti di filiera per il settore forestale è stato caratterizzato da una vasta partecipazione, con un *overbooking* di circa 50 milioni di euro. Lo scorrimento delle graduatorie menzionate avverrà nel rispetto delle condizionalità tipicamente richieste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Conseguentemente, i progetti potranno essere finanziati, se in linea con gli obblighi di contributo al *target* individuato dalla Commissione europea, nonché con quelli previsti in materia dal secondo cui gli interventi del PNRR nazionali non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente. A tale riguardo, preciso che il Ministero è in attesa dello schema di *operational gli accordi operativi subordinati alla decisione europea, che permetteranno di individuare correttamente tutti i contenuti necessari per la menzionata convenzione tra il Ministero e l'Ismea, punto di partenza di successive attività di scorrimento delle graduatorie. Inoltre, sono funzionali alla puntuale individuazione del meccanismo di verifica di *milestone* e *target*, nonché del rispetto delle diverse condizionalità specifiche connesse alla misura e quindi all'identificazione e declinazione delle condizionalità da applicare, che non potranno essere quelle connesse al PNRR. In merito alla necessità di ottenere ulteriori fondi, segnalo che con la rimodulazione del PNNR le risorse a disposizione del settore agricolo sono sostanzialmente raddoppiate, passando da 3,6 miliardi a 6,4 miliardi. Se si considerano anche quelle del PNC, cioè del Piano nazionale complementare, si arriva a circa 8 miliardi. Si tratta adesso di concretizzare questi investimenti, fermo restando che, qualora residuassero iniziative non finanziate, verranno attivate tutte le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse.

Volevo porre all'attenzione del Sottosegretario il tema cruciale che riguarda come intendiamo in tempi rapidi sostenere la filiera dell'agroalimentare italiano, perché sicuramente ci rendiamo tutti conto che abbiamo una grandissima opportunità. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta, per una delle filiere più importanti del *made in Italy* italiano, una grande occasione per produrre innovazione, generare lavoro, crescita e sviluppo economico. La nostra preoccupazione resta nei tempi. Questa interrogazione ha come finalità quella di cercare di stimolare lo scorrimento delle graduatorie e la necessità di costruire nel Governo una visione autentica di filiera, che non dimentichi le intere componenti della filiera. Non ci sono solo le grandi imprese; dietro una grande impresa, soprattutto nell'agroalimentare, c'è una moltitudine di piccole e medie imprese che vanno tenute dentro i processi di innovazione che il Piano nazionale di ripresa e resilienza può determinare. signor Sottosegretario, era orientata a porre all'attenzione del Governo il tema dei tempi, quello di una visione industriale di sviluppo economico del Paese e quello del sostegno alla competitività economica di una quantità innumerevole di imprese, che, se non lasciate da sole, possono rappresentare una condizione vera di sviluppo economico e di crescita. Sa quanto noi, signor Sottosegretario, che l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è decisiva anche per sostenere la crescita e la pur bassa crescita che oggi viene individuata è tutta legata ai tempi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ci raccomandiamo a lei, innanzitutto, affinché si proceda rapidamente e si assuma una visione coerente dello sviluppo economico del nostro Paese. Serve una visione autentica dello sviluppo industriale nella filiera dell'agroalimentare, serve un pensiero autentico di filiera, che tenga insieme grandi e piccole imprese che rappresentano un potenziale enorme di crescita e di sviluppo economico di un comparto decisivo anche per generare nuova occupazione e - aggiungo - anche livelli occupazionali adeguati, con salari giusti e dignitosi. Quindi, ci raccomandiamo che i tempi siano celeri e che si proceda con più velocità rispetto a quello che si sta facendo. Il tempo dell'orientamento è finito, ora servono le risorse per consentire alle imprese di crescere in innovazione e di agganciare le filiere più importanti dello sviluppo, anche nella dimensione europea. Per cui monitoreremo i tempi e la invitiamo a tenere conto del fatto che i tempi saranno decisivi anche per lo sviluppo economico del nostro Paese.

il 17 luglio 2023 l'associazione ambientalista Mareamico, delegazione di Agrigento, indirizzava alla Capitaneria di Porto Empedocle un esposto in merito alla rottura della condotta sottomarina di allontanamento in mare di reflui urbani, sita in località Canne, nel Comune di Siculiana, in provincia di Agrigento. In pari data la Capitaneria di porto disponeva l'uscita di un proprio mezzo nautico con due tecnici dell'ARPA Agrigento per il sopralluogo e campionamento di acque di mare nello specchio acqueo interessato dallo sversamento di reflui fognari. L'ARPA segnalava la perdita di acque reflue dalla condotta di allontanamento a circa 50 metri dalla battigia, che aveva generato una chiazza surnatante marrone, estesa su una superficie marina di diametro circa pari a 50 metri. Nella stessa giornata l'AICA (Azienda idrica comuni agrigentini) preannunciava l'intervento in regime di urgenza di una ditta specializzata, al fine di verificare l'entità e la natura dell'evento occorso, per la risoluzione della criticità riscontrata. Il 19 luglio 2023 sempre l'AICA partecipava alla Capitaneria di Porto Empedocle e, per competenza, anche al sindaco del Comune di Siculiana, all'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e al dipartimento dell'ambiente e strutture territoriali di Agrigento e Caltanissetta i risultati della verifica effettuata dalla stessa ditta, rappresentando che a circa 35 metri dalla costa, dove termina la parte interrata della condotta, risultava mancante, per cause non note, un tratto di 15 metri. Il Reparto ambientale marino del Corpo della Capitaneria di porto avviava un intervento urgente volto alla sostituzione di circa 40 metri della condotta sottomarina riguardante il tratto mancante e quello adiacente, connotato da segni di vetustà e pregresse riparazioni. Ancora in seguito, il 16 agosto 2023, l'ARPA Sicilia comunicava gli esiti analitici relativi ai campioni di acqua di mare prelevati il 17 luglio 2023, evidenziando concentrazioni elevate di ione ammonio ed escherichia escherichia coli, di cui il RAM notiziava la procura della Repubblica territoriale competente. Infine, in data 18 agosto 2023, l'AICA comunicava il ripristino della funzionalità della condotta, preannunciando un nuovo intervento dei sommozzatori per la verifica di un giunto di collegamento posto a circa 130 metri dalla linea di costa. Tanto specificato, premesso che il MASE è costantemente impegnato a vigilare, intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche inerenti al settore fognario-depurativo, si sottolinea che gli scarichi delle pubbliche fognature con condotte sottomarine sono regolamentati con legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, rispetto ai cui articoli 8 e 11, attinenti ai livelli di depurazione e ai relativi limiti di accettabilità, il RAM non segnala difformità. Al riguardo si rammenta altresì che la depurazione, e conseguentemente la gestione degli impianti, rientra nel processo verticale del servizio idrico integrato e che l'articolo 149, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2006 affida agli enti di governo d'ambito la ricognizione delle infrastrutture, la pianificazione degli interventi, nonché l'elaborazione del relativo piano economico-finanziario. Inoltre, la competenza primaria in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione, a mente del decreto-legge n. 116 del 2008, è in capo al Ministero della salute. Regioni e Province autonome, seguendo la normativa di settore, classificano le acque di balneazione secondo una qualità scarsa, sufficiente, buona ed eccellente. Ove la classe sia eccellente, il profilo deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione diviene buona, sufficiente o scarsa. Dal portale delle acque gestito dal Ministero della salute emerge che i siti di balneazione Foce Vallone e Torre Salsa, nel Comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, sono in classe eccellente.

caro Sottosegretario, che stiamo parlando di un evento che è avvenuto all'interno di una riserva naturale orientata di grande interesse, in pieno luglio. Come ha ben detto lei, anche a seguito delle indagini dei vari soggetti coinvolti, dal reparto ambientale marino della Guardia costiera, dall'ARPA, dal nucleo dei carabinieri specializzati in tutela ambientale,

è oggetto dell'ultima procedura di infrazione. Come ben sappiamo, l'Italia, e la Sicilia in particolare, sono soggette a ben quattro procedure di infrazione, di cui tre già con condanna definitiva.

della frazione marina di Siculiana. Pertanto, mi aspettavo anche di ricevere informazioni, magari tramite le interlocuzioni tra il Ministero dell'ambiente e la struttura commissariale, che proprio la rete di collettamento e fognaria della frazione marina di Siculiana è quella imputata ed inserita nella procedura di infrazione. Attualmente, la parte dei reflui fognari di quella frazione viene solamente in parte intercettata. Si fa una mera grigliatura. Si parla di attività preliminari, ma, in buona sostanza, vi è una grigliatura, l'acqua viene rimandata all'uscita dal depuratore di Siculiana, reimmessa in condotta tal quale ed inviata a mare.

di tutto il ciclo delle acque, si è insediata da poco, a seguito anche delle vicende giudiziarie legate a Girgenti Acque. Però, nella sostanza, quello che si chiede, oltre alla massima attenzione, è di avere ulteriori informazioni in relazione alla procedura di infrazione e di sapere quando riusciremo a far depurare i reflui prodotti da questa frazione. Ribadisco questi reflui vengono immessi direttamente in mare, tal quali, in una riserva naturale orientata. La riserva naturale di Torre Salsa è un gioiello riconosciuto a livello internazionale. E noi cosa facciamo? scarichiamo parti di reflui non trattati? Questo non è ammissibile e, non a caso, è in corso una procedura di infrazione. Ricordo all'Assemblea e ai colleghi, che noi paghiamo 165.000 euro al giorno per una delle quattro procedure di infrazione, che ci costano 60 milioni di euro l'anno.

e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo al quesito posto sulla base degli elementi forniti dalla Provincia autonoma di Trento. infatti, che la gestione della strada statale 240 di Loppio e Val di Ledro è passata, in seguito al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, dalla società Anas allo stesso ente provinciale. In premessa, la Provincia di Trento ha rappresentato che svolge una regolare attività di monitoraggio e manutenzione delle due gallerie. In riferimento alla galleria Agnese, il monitoraggio ha evidenziato che l'ammasso roccioso, che questa galleria attraversa non presenta particolari criticità. Per quanto riguarda la galleria Dom, questa è stata oggetto di un attento monitoraggio geologico e strutturale da parte della Provincia a partire dal 2011, in esito al quale, nel mese di febbraio 2023, è stato redatto un documento preliminare di progettazione per la realizzazione di un rinforzo strutturale tramite chiusura alla base della volta, drenaggi, chiodature e rinforzo strutturale della volta. Inoltre nell'ultimo quinquennio, oltre agli ordinari interventi di manutenzione e controllo degli elementi costitutivi del tunnel, sono state realizzate diverse attività, tra le quali: il rifacimento a più riprese della segnaletica orizzontale per l'intera galleria, la verifica dell'efficienza e la pulizia delle opere di drenaggio presenti all'interno del tunnel; la manutenzione straordinaria della pavimentazione bituminosa nei tratti più ammalorati; le verifiche periodiche di efficienza degli impianti tecnologici e la sostituzione dei componenti guasti o usurati; la verifica dello stato di sollecitazione del rivestimento in calcestruzzo della galleria in alcuni punti. In merito agli specifici interventi di messa in sicurezza posti in essere in seguito al distacco di una porzione del rivestimento in calcestruzzo della galleria Dom, avvenuta il 5 novembre 2023, in prossimità del chilometro 20+200 circa della strada statale 240, si rappresenta che il personale addetto alla manutenzione dell'arteria viaria, in collaborazione con i geologi della Provincia, ha immediatamente avviato, con procedura di somma urgenza i rilievi e le attività per la messa in sicurezza del tunnel nel tratto interessato dalla frana. Sulla base dei rilievi preliminari svolti, il successivo 7 novembre sono stati intrapresi i lavori di prima fase finalizzati alla stabilizzazione del rivestimento in calcestruzzo mediante l'esecuzione di una bullonatura radiale con barre in acciaio della lunghezza di 6 metri per un tratto di galleria di circa 21 metri a cavallo del tratto interessato dal distacco. Già a partire dal 13 novembre 2023, ultimata la bullonatura del tratto in corrispondenza della porzione interessata dal distacco, è stato possibile ripristinare la circolazione all'interno della galleria nella fascia oraria 6-22, a senso unico alternato con impianto semaforico, con la prosecuzione dei lavori esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6. In riferimento alle soluzioni alternative per far fronte ai disagi maturati maturati dal crollo, le interlocuzioni con le amministrazioni sono state costanti e proficue fin dalla fase iniziale dell'evento e con le stesse sono state valutate le diverse opzioni, tra le quali quelle citate dai senatori interroganti. In merito all'utilizzo del corridoio San Giacomo, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Riva del Garda, è stata valutata l'opzione di utilizzarlo come collegamento alternativo tra la Val di Ledro e l'Alto Garda. Tenuto conto delle sue caratteristiche geometriche e di tracciato, tale soluzione è stata ritenuta praticabile esclusivamente per i mezzi di soccorso quali ambulanze e mezzi leggeri dei Vigili del fuoco. A tal fine è stato definito uno specifico protocollo d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti. Per quanto attiene alla proposta di attivare un bus navetta attraverso lo stesso corridoio, va sottolineato che già a partire dal 13 novembre 2023 è stato ripristinato il collegamento viario tra l'Alto Garda e la Val di Ledro nella fascia oraria 6-22 e che i lavori di consolidamento della galleria Dom sono stati limitati alla fascia oraria notturna dalle 22 alle 6. Inoltre, le verifiche tecniche eseguite di concerto con l'amministrazione comunale di Riva del Garda hanno evidenziato che tale collegamento non era praticabile in quanto non presentava adeguati margini di sicurezza per le caratteristiche geometriche di tracciato. I lavori sono proseguiti con una temporanea sospensione, disposta su richiesta delle amministrazioni locali e degli operatori economici dell'Alto Garda e della Val di Ledro, per consentire la libera circolazione nella galleria Dom anche in orario notturno anche in orario notturno dal 22 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024, in corrispondenza del periodo di festività. L'ultimazione degli interventi per il consolidamento dei rivestimenti del tunnel era stata prevista pertanto entro le prime era stata prevista pertanto entro le prime due settimane di febbraio 2024. Nel dettaglio si è trattato di ricostruire la porzione del rivestimento crollato mediante posa in opera a strati successivi di calcestruzzo armato, previa pulizia e regolarizzazione delle superfici a contatto con la parete rocciosa, nonché di rinforzare il rivestimento della galleria attraverso la posa di centine formate da profili metallici, alle quali è stato applicato il calcestruzzo per ripristinare l'originale sagoma. L'intero sviluppo della volta è stato poi rivestito con una lamiera in acciaio inossidabile, in modo da ripristinare l'impermeabilizzazione del tunnel. A completamento dei lavori sono state potenziate le opere per il drenaggio e il convogliamento delle acque, al fine di prevenire riversamenti e ristagni sulla strada. Da segnalare, infine, che per consentire il ripristino e il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo, si è reso necessario il preventivo spostamento provvisorio degli impianti tecnologici a servizio della galleria, che sono stati riposizionati al termine dei lavori. Il cronoprogramma dei lavori indicati è stato pienamente rispettato e lo scorso 16 febbraio la galleria Dom è stata riaperta al pubblico garantendo il ripristino della piena funzionalità del tunnel stradale, restituendo al territorio questa importante arteria.

problema, tuttavia, non si risolve soltanto elencando i provvedimenti assunti, perché, come ho cercato di dire nell'interrogazione, si tratta di una situazione molto particolare di una valle isolata rispetto al resto del territorio e accessibile soltanto attraverso percorsi geologicamente a rischio. Non a caso, nella fase intercorrente tra la presentazione dell'interrogazione e la risposta di oggi è franato un altro tratto della strada statale SS240, in corrispondenza del lago di Ledro, a testimoniare i i cambiamenti climatici in atto, abbinati al fatto che gli inverni sono miti e quindi l'effetto gelo-disgelo, che, come sappiamo, molto spesso è responsabile di disgregazioni della roccia,

spinge il soffitto della galleria e lo fa cedere, non potremo continuare a interrompere i flussi di traffico e quindi i collegamenti tra una valle e il resto del territorio, su una strada percorsa ogni

l'alternativa viene giudicata non praticabile, quindi adesso risistemiamo la galleria e ci auguriamo che Dio ce la mandi buona. Non so se sia davvero la soluzione finale, ma auspico che lo sia, perché chiaramente non ho nessun interesse che ci siano ulteriori incidenti. La mia paura, purtroppo, è che ce ne potranno essere.

alle quali risponderanno il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Presidente, signor Ministro, più volte in questa legislatura abbiamo parlato in quest'Aula con lei di misure che aiutino a combattere l'inquinamento, le emissioni di gas serra e la promozione e diffusione delle fonti rinnovabili. In questo ambito il suo Ministero ha recentemente pubblicato il cosiddetto decreto agrivoltaico, in vigore dal 14 febbraio. Il decreto intende promuovere la realizzazione di agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia elettrica pulita. Da una parte le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento e una tariffa incentivante sull'energia immessa in rete. Sicuramente questa coesistenza tra produzione agricola e produzione di energia elettrica consentirà di garantire risparmi e vantaggi all'attività primaria delle stesse aziende agricole. Le chiediamo quindi, signor Ministro, quali sono le caratteristiche innovative, gli investimenti previsti, la potenza che prevedete verrà installata in Italia e i benefici attesi dall'agrivoltaico.

Il decreto ministeriale cosiddetto agrivoltaico rappresenta un tassello della grande sfida volta a far coesistere l'eccellenza agricola con soluzioni energetiche sostenibili. Assieme alle comunità energetiche questo è probabilmente uno dei provvedimenti più qualificanti per cambiare dal territorio il paradigma energetico del nostro Paese e guardare al futuro. Il decreto si pone l'obiettivo di potenza installata complessiva pari almeno a 1,4 gigawatt e per una produzione indicativa di almeno 1.300 gigawatt entro il 2026. In questo contesto, il decreto cosiddetto agrivoltaico promuove soluzioni costruttive innovative, con la possibilità di coesistenza di più usi del suolo e con benefici aggiuntivi legati alla compatibilità della produzione di energia con le attività agricole, anche al fine del recupero dei terreni all'uso produttivo. La misura prevede un contributo in conto capitale, nel limite del 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, finanziato con oltre un miliardo di euro di risorse PNRR, cui si abbina un incentivo a tariffa della durata di vent'anni applicato alla produzione di energia elettrica netta messa in rete. Le procedure di registro previste per complessivi 300 megawatt sono riservate ad impianti di potenza fino a un megawatt realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni; mentre le procedure competitive, per complessivi 740 megawatt, sono dedicate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni o associazioni temporanee di impresa con almeno un imprenditore agricolo. Un altro punto cardine del decreto è il sistema di monitoraggio dell'attività agricola sottostante per valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero di fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture. In conclusione, la misura vuol essere un volano per l'innovazione del settore e per gli obiettivi fissati per il 2030 dal Piano nazionale integrato energia e clima, in termini di quota totale di energia da rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, in un'ottica di sostenibilità ambientale, favorendo altresì la resilienza anche in chiave economica delle aziende agricole coinvolte. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Rosso, Signor Presidente, sono particolarmente soddisfatto della risposta del Ministro e mi complimento con lui per la capacità di una visione rivolta al futuro. Gli americani direbbero che è un decreto *win-win*, ovvero dove vincono tutti. Vince il mondo dell'agricoltura che, attraverso soluzioni costruttive e innovative, permetterà la coesistenza di più usi del suolo, il recupero di terreni all'uso produttivo, il recupero della fertilità del suolo e la resilienza delle colture ai cambiamenti climatici, ma vince anche l'ambiente, Ministro, e cioè vincono i cittadini, che avranno più risparmio idrico e una riduzione dell'inquinamento grazie all'aumento di produzione di energia elettrica pulita. Questa misura agrivoltaica conferma ulteriormente la linea della maggioranza di centrodestra e di Forza Italia in merito agli obiettivi di decarbonizzazione, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e indipendenza energetica. Quindi, bravo ministro Pichetto, questo Governo dimostra che la tutela dell'ambiente non è solo ad appannaggio delle sinistre; anzi, a sinistra c'è chi si riempie sempre la bocca di proclami, ma i fatti li fa il Governo di centrodestra.

finestra") *(IV-C-RE)*. Ministro Urso, forse per limiti personali, noi non riusciamo a comprendere quale sia la linea di politica industriale di questo Governo. Vi faccio qualche esempio. nel mese di agosto si è molto lamentato - e aveva ragione - sul caro dei biglietti aerei, tanto da dire che sarebbe intervenuto su Ryanair, cosa che ha fatto, salvo poi dover tornare indietro, anche perché l'Unione europea le ha ricordato che quello sarebbe stato un elemento contro la concorrenza; oppure dire che avreste messo un limite al prezzo del gasolio, salvo poi dimenticarsi nella legge di bilancio di non aumentare quelle diminuzioni delle accise che erano intervenute durante il Governo Draghi. quando c'è una crisi industriale, la sensazione è sempre che la sua prima dichiarazione sia di intervento dello Stato nell'ambito industriale, salvo poi un po' un po' di ravvedimenti. Le faccio un esempio che mi tocca molto da vicino, perché sono di Torino: quanto a Stellantis e alla crisi dell'auto, lei ha annunciato anche la disponibilità dello Stato di entrare in Stellantis, che sarebbe stata la prima volta in Italia. Lei mi dirà che la FIAT, la vecchia FIAT, ha ottenuto tanti soldi dagli italiani: questo è vero, vero, ma è sempre stata un'impresa privata. Veniamo a Ilva. In questo periodo abbiamo il decreto Ilva in 9a Commissione che evolve ogni settimana, però cos'è che ci preoccupa? Lei aveva detto che andava abbastanza bene la situazione, tanto da aver messo addirittura dei soldi pubblici, salvo poi doversi ravvedere di fronte alle manifestazioni di chi fa parte dell'indotto, che non ha ricevuto i soldi da parte dell'ex Ilva, dai sindaci di centrodestra e di centrosinistra. Noi abbiamo audito tutti i Presidenti e casualmente, tranne un Presidente di centrosinistra (Emiliano), gli altri due centrodestra) hanno manifestato la preoccupazione per l'occupazione, per l'indotto e per il fatto che il nostro Paese non può fare a meno dell'acciaio. Arrivo alla domanda: che cosa farete su Ilva? Noi non l'abbiamo capito. L'abbiamo avuta anche in audizione e mi è sembrata di nuovo un'interlocuzione sul presente piuttosto che una prospettiva sul futuro, posto che chi le parla non ha alcuna nostalgia di ArcelorMittal. Nel momento in cui si toglie toglie un soggetto privato, però, cosa vuol dire? Si va verso la nazionalizzazione dell'acciaio o si trova un altro acquirente privato? E se sì, con quali condizioni? Ad esempio, lo scudo penale tolto in maniera improvvida dal Governo giallo-verde

e rispondo che non è vero - come affermato - che è stata ritirata la misura sul caro voli. Anzi, è stata resa più efficace, nel confronto con il Parlamento, rafforzando i poteri istruttori e sanzionatori dell'Autorità per la concorrenza. Da ciò è già conseguito un primo provvedimento dell'Autorità, che ha avallato la linea del Governo, e anche l'Europa ci ha dato ragione, aprendo a sua volta un *focus* sul caro voli. Nell'interrogazione poi si parlava del caro taxi e non è vero che è stata fatta retromarcia in materia. Anzi, sempre con il decreto-legge *asset*, siamo intervenuti in maniera efficace a riformare il settore, laddove altri tre Governi avevano clamorosamente fallito: Monti nel 2011, Renzi nel 2016 e Draghi nel 2022, ritirando, loro sì, le riforme presentate in Parlamento. Infatti, con la nostra riforma, alcuni Comuni come Milano, Firenze e Bologna hanno già utilizzato la nuova efficace normativa per accrescere il numero di taxi in servizio. L'interrogazione si riferisce anche all'inflazione. Bene, proprio questa mattina i dati Eurostat ci dicono che l'Italia e la Danimarca sono i due Paesi in Europa in cui l'inflazione cresce meno, con tassi annuali dello 0,9 per cento, a fronte della media dell'eurozona di tre volte superiore (2,8). Quando arrivammo al Governo, il tasso di crescita annuale era dell'11,8; oggi è la più bassa d'Europa. In merito poi all'interrogazione che dice che noi utilizziamo troppo spesso lo strumento della *golden power*, faccio notare che, su 477 procedimenti di competenza del Ministero, è stato fatto ricorso alle prescrizioni in 26 casi (prescrizioni significa condizionamenti, liberando l'investimento a condizione di salvaguardare tecnologia, produttività e occupazione). Solo in un caso è stato fatto ricorso al potere di veto; solo in un caso su 477. riguardava nello specifico un investimento riconducibile a un'operazione russa, a cui peraltro è collegato proprio un soggetto molto vicino alla forza politica che oggi mi rivolge il quesito. Se vi riferite a questa operazione, sappiate che noi non subordiniamo gli interessi nazionali agli interessi privati, mai. In merito all'ex Ilva di Taranto, abbiamo nominato in poche ore il commissario, da tutti riconosciuto come la migliore scelta possibile (dai sindacati, tutti i sindacati, come da tutte le associazioni che rappresentano l'impresa), con l'obiettivo immediato di mettere in salvaguardia lo stabilimento, rilanciare la produzione, attivare il *revamping* degli altoforni, mettere in sicurezza gli impianti e i lavoratori; ciò al fine di realizzare le migliori condizioni per accogliere i nuovi investitori e contribuire al rilancio della siderurgia italiana.

lo dica alla sua collega Santanchè, che non più tardi della scorsa settimana ha fatto un bellissimo *tweet* con cui denunciava la situazione drammatica dei taxi in Italia, come se non facesse parte di questo Governo. Per quanto riguarda la *golden power*, le posso soltanto suggerire di scrivere anche il regolamento sulla *golden power* dell'idroelettrico. Avrebbero dovuto farlo entro sessanta giorni dalla concorrenza, ma questo non è ancora avvenuto, con il rischio di regalare, questo sì, a stranieri, l'acqua e l'energia.

per i privati che verranno a investire in Italia, di non essere sottoposti a quanto hanno vissuto già gli altri privati, cioè alla chiusura di forni da parte della magistratura e ai continui *stop* della produzione che di fatto sono avvenuti? oggi abbiamo un commissariamento, ma sapete benissimo che i soggetti dell'indotto hanno una paura, fondamentale e fondata, dati gli emendamenti che avete presentato. La paura è quella di non ottenere quanto loro hanno già dato e prodotto, ma non hanno ricevuto indietro in soldi. Il vostro emendamento prevede un limite

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale - che, lo ricordo, sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti - e alla quale partecipa anche l'Unione europea. La Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà su tutto su tutto il territorio nazionale. Per lo sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, ai quali saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane. Il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà il 13 marzo prossimo a Verona. Il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei Ministri del G7, avente ad oggetto industria, tecnologia e digitale, cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il *summit* sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale. In questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici. Le chiedo, signor Ministro, quali sono gli obiettivi che intende perseguire con la sua presidenza: di quali proposte si fa portatrice l'Italia e cosa si attende dagli incontri menzionati nella premessa che ho fatto?

Non a caso abbiamo deciso di focalizzarla sui temi più sfidanti per le imprese, in un'epoca di grandi cambiamenti tecnologici e geopolitici. Alla vigilia di tale riunione ci sarà anche una conferenza dei portatori di interesse con i CEO delle più importanti aziende dei sette Paesi. Cercheremo di valutare come far convergere le nostre politiche industriali in questa delicata e difficile fase dell'agenda internazionale, in cui conflitti sempre più gravi sono intorno alla nostra Europa, con nuovi rischi per gli assetti geoeconomici globali.

proprio perché siamo convinti, oggi più che mai, che serva una chiara visione strategica di politica industriale condivisa con i nostri alleati. Sono stati invitati a partecipare anche Corea del Sud, Emirati Arabi e Ucraina, per il contributo importante che possono dare al confronto, segnale politico significativo in aree strategiche anche per la sicurezza e lo sviluppo economico. L'Italia si farà portatrice di tre filoni. è l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale, con l'obiettivo di assicurare che lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie siano funzionali a un incremento tangibile della produttività e della competitività dei nostri sistemi industriali. la sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti, con l'obiettivo di realizzare un coordinamento sui semiconduttori per ridurre la dipendenza da Paesi terzi e realizzare canali di connettività spaziali e sottomarini in sicurezza. occorre sviluppare digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un *focus* sull'Africa, in linea con il Piano Mattei, affinché anche quei Paesi beneficino delle potenzialità dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. L'Italia è protagonista, finalmente, con una visione strategica, che coniuga interesse nazionale con la tutela dei valori fondamentali di libertà e la necessità di uno sviluppo sostenibile.

Signor Presidente, oggi sottopongo all'attenzione del ministro della salute Orazio Schillaci una questione che mi sta molto a cuore, perché riguarda la sanità pubblica e quindi, di riflesso, la salute dei nostri cittadini. Viviamo in un'epoca in cui la digitalizzazione è un processo che riguarda a trecentosessanta gradi le nostre vite. Il digitale e dunque le nuove tecnologie possono svolgere potenzialmente un importante ruolo anche e soprattutto in ambito sanitario. Questo Governo si è impegnato da subito su questo fronte. Ricordo l'impegno dell'Esecutivo e in modo particolare il suo, signor Ministro, per superare l'*impasse* del fascicolo sanitario elettronico, a breve basterà accedere a questo dispositivo per conoscere tutta la storia clinica di un assistito. Dobbiamo proseguire con forza in questa direzione. In linea con la prospettiva di creare una sanità formato 5.0, quindi completamente digitalizzata, ci sono le risorse, ad esempio quelle europee previste dal PNRR, in modo particolare con riferimento alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione delle strutture ospedaliere. In questo contesto la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, ad esempio, rivestono un ruolo fondamentale anche, ma non solo, nel sistema di raccolta e analisi dei dati. Il dato oggi dei dati. Il dato oggi - come ben sappiamo - è una materia fondamentale e lo è ancor di più se si intende utilizzarlo in maniera strategica per definire una programmazione sanitaria efficace, per promuovere la ricerca e, soprattutto, per definire i giusti ed efficaci percorsi per la prevenzione delle malattie. Se è vero che tanto lavoro è stato fatto, è certamente altrettanto vero che tanto lavoro resta ancora da fare. La sfida di una sanità digitale e sostenibile - come ha detto lei più volte, signor Ministro - è cambiare completamente il paradigma per fortificare il nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo cambiare modello. Al ministro Schillaci chiediamo, come Gruppo UDC-Coraggio Italia-MAIE, quali siano state le azioni finora intraprese dal Governo per sostenere la transizione digitale del Servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo dall'Esecutivo per sfruttare le risorse del PNRR nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il Servizio sanitario a domicilio del paziente; una sanità digitale intesa anche come sinonimo di sanità sostenibile per portare a una riduzione degli accessi impropri, quindi più efficiente ed efficace, e per dare più servizi ai cittadini in tempi sempre più veloci e, più in generale, mettendo in campo tutte le possibili soluzioni volte a migliorare la vita degli italiani.

che vede il domicilio come primo luogo di cura, con particolare riferimento ai pazienti cronici e fragili, in coerenza con il quadro normativo della riforma dell'assistenza territoriale, nell'ambito di un progetto unitario di riforma dell'assistenza del territorio con l'integrazione del digitale. In questo contesto, la sanità digitale rappresenta uno strumento con cui raggiungere tale obiettivo. Si stanno portando avanti diverse politiche e investimenti finalizzati a promuovere l'avanzamento tecnologico e digitale del nostro Sistema sanitario nazionale. A tale scopo sono stati destinati circa 3 miliardi di euro del finanziamento europeo NextGenerationEU. Nello specifico, 1,3 miliardi sono dedicati al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, 1,5 miliardi alla telemedicina e circa 200 milioni di euro per investimenti a creare piattaforme informatiche nazionali, sviluppo e adozione di nuovi flussi informativi nazionali e strumenti digitali di *governance.* L'investimento relativo al fascicolo sanitario elettronico, in particolare, ha l'obiettivo di garantire la completa diffusione sul territorio nazionale e di rafforzarne l'utilizzo in ottica di monitoraggio e programmazione dei servizi sanitari. L'investimento prevede un processo di armonizzazione della raccolta dei dati che permette di migliorare la qualità degli stessi e la creazione di un ecosistema di dati sanitari. Per quanto riguarda la telemedicina, nel 2023 è stata realizzata dall'Agenzia la piattaforma nazionale di telemedicina con funzioni di governo e monitoraggio delle prestazioni sanitarie. Questa piattaforma permette di armonizzare a livello nazionale codifiche *standard*, implementare e gestire i processi, monitorare l'attuazione e la misurazione dei reali benefici i risultati conseguiti. All'interno dell'investimento è in corso, inoltre, la realizzazione delle infrastrutture regionali di telemedicina, attraverso le quali avverrà l'erogazione dei servizi sanitari da remoto. Consapevoli dell'importanza del governo delle attività di digitalizzazione e dell'impatto di quest'ultime sull'organizzazione dei servizi sanitari, lo scorso anno è stata istituita presso l'Agenas l'Agenzia nazionale di sanità digitale, con il compito di definire, aggiornare e diffondere documenti di indirizzo e linee guida prescrittivi per Regioni e Province autonome. altresì che mediante i fondi del PNRR viene finanziata la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto delle cure primarie, per aiutare il medico nelle attività di cura e a snellire il carico amministrativo e organizzativo. Infine, nell'interrogazione del senatore De Poli spicca una parola importante che guida il nostro mandato: «sostenibilità». Il cambiamento degli scenari e degli stili di vita ci chiede di ripensare il Servizio sanitario nazionale per renderlo equo per tutti e per davvero. Innovazione e digitalizzazione saranno la chiave di un nuovo modello basato sulla prevenzione e sull'anticipazione delle patologie. Questo Ministero sarà a fianco di tutte le Regioni che stanno lavorando per rendere le strutture più efficienti ed efficaci. Allo stesso tempo, non mancheremo di vigilare su sprechi e inadeguatezze.

non solo della sanità, ma in tutto il contesto pubblico della nostra Nazione. Proprio per questo motivo uso una parola forse non consueta, ma che mi piace in questa sede: bravo, signor Ministro, perché la salute di ognuno di noi è il bene più grande che abbiamo.

Signor Presidente, signor Ministro, secondo un'inchiesta pubblicata dalla «Kronen Zeitung», il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto *toe trimming*. Si tratta della bruciatura della punta delle zampe di tacchini appena nati che, secondo tutti gli studi, è fonte di enorme sofferenza per gli animali. Tale procedura viene effettuata solo per massimizzare i profitti, per evitare che i tacchini ammassati negli allevamenti intensivi si graffino a vicenda, compromettendo la qualità delle carni. In Austria, dove la pratica è vietata, il *toe trimming* degli allevatori italiani solleva da tempo numerose reazioni. Le locali organizzazioni degli allevatori chiedono che gli esercizi commerciali eliminino dai loro scaffali prodotti italiani o che, in alternativa, non vengano esposti accanto a quegli austriaci, perché le carni austriache sono prodotte garantendo meno sofferenze per gli animali e per questo possono avere prezzi più alti. Considerato che il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva europea sulla protezione degli animali negli allevamenti,

Inoltre l'inchiesta giornalistica rischia di compromettere un comparto che fa del *made in Italy* un sinonimo di qualità e che invece potrebbe essere associato a pratiche che causano sofferenze agli animali. Si chiede pertanto di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del *toe trimming* all'interno degli allevamenti di tacchini, se può fornire informazioni sul numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano e se non intenda introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti di tacchini e vietare esplicitamente la pratica del *toe trimming.*

Questo principio ha influenzato anche la legislazione comunitaria, portando non solo ad emanare numerose forme finalizzate alla protezione degli animali, ma anche a riconoscere la necessità di tener conto, nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Ciò premesso, con riferimento alla troncatura delle unghie delle tacchine di un giorno di vita, mi preme rappresentare che nel 2019 il Ministero della salute, acquisito il competente parere del Centro di referenza nazionale per il benessere animale, ha indicato agli assessorati alla sanità la possibilità di ricorrere al procedimento del *microwave claw processor* (MCP), avvalendosi di personale qualificato e adeguatamente formato allo scopo. Detto procedimento ha aggiornato la previgente pratica della troncatura delle unghie nell'ottica di ridurre al minimo lo stato di sofferenza. Nello specifico. il parere reso dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale ha consentito di rilevare che il procedimento MCP, meglio tollerato rispetto ad altre tecniche tradizionali, porta ad un'incidenza ridotta di graffi e lacerazioni cutanee, tipiche delle tacchine femmine, che tendono a saltare sopra agli altri animali nella fase di allevamento e di trasporto, causando sofferenze ed effetti negativi sulla salute animale. Si è potuto accertare pertanto un riscontro positivo a favore della metodica MCP nel rapporto tra beneficio e danno rispetto al benessere degli animali allevati. Con riferimento alla richiesta di informazioni riguardo al numero degli allevamenti presenti sul territorio nazionale, rappresento che alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica al 31 dicembre scorso risulta che in Italia sono registrati 795 allevamenti di tacchini da ingrasso, per un totale di 9.082.322 capi, e 53 allevamenti di tacchini da riproduzione, per un totale di 427.581 capi.

con sistemi innovativi digitalizzati quale quello messo a punto dal predetto centro di referenze, denominato *classyfarm*, per avere ulteriori elementi di valutazione nell'ottica di assicurare comunque agli animali allevati condizioni di benessere sostenibili nell'ambito degli *standard* definiti dall'Unione europea.

mi dice che va fatta in un modo che fa soffrire il meno possibile gli animali. Il fatto però che in altri Stati che hanno uno *standard* di tutela degli animali molto più elevato, come l'Austria, sia vietato dimostra che non è una pratica che non procura tante sofferenze agli animali. La pregherei di valutare se non sia necessario introdurre anche in Italia il divieto di questa pratica e aumentare gli spazi e la superficie per i tacchini, che porterebbe allo stesso risultato senza arrecare atroci sofferenze agli animali.

per contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l'erogazione di ortesi, protesi, ausili e dispositivi di tecnologia avanzata, funzionali anche all'attività sportiva amatoriale. occorreva un decreto ministeriale, chiaramente del Ministro della salute, di concerto con il MEF e d'intesa con le Regioni;

i suoi effetti risultano deludenti e la misura prevista è sostanzialmente inapplicata per l'assenza d'informazione delle preposte strutture del Servizio sanitario nazionale. Mi arrivano sollecitazioni e frequenti segnalazioni di persone con disabilità che fanno richiesta, che hanno tutti i requisiti, ma si

non si capisce esattamente dove si sia impuntato il carro, per così dire. Gliela faccio breve: le chiedo di sapere esattamente, Ministro, cos'ha fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura e, in particolare, se ha modo di relazionare su quante e quali Regioni hanno di fatto ripartito questo fondo e ne hanno disciplinato l'utilizzo. Questa sperimentazione serviva per dimostrare la reale esigenza, urgente e sentita,

n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, adottando il decreto ministeriale 22 agosto 2022, nel quale sono stati definiti tetti di spesa per ciascuna Regione che accede al Fondo sanitario nazionale con i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori. L'articolo 3 del suddetto decreto, in particolare, ripartisce tra le Regioni il finanziamento pari a 5 milioni per l'erogazione delle protesi e degli ausili. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costituisce di per sé una comunicazione da parte del Ministero a tutte le Regioni e ai soggetti interessati, senza che si debbano a tal riguardo attuare ulteriori adempimenti informativi. Per quel che concerne il monitoraggio, si rileva che l'articolo 2 prevede che il modulo di prescrizione dei dispositivi oggetto della sperimentazione indichi le modalità di *follow up* del programma, nonché la verifica degli esiti. Tale *follow up* dev'essere effettuato dal medico specialista responsabile della prescrizione. Le aziende sanitarie erogatrici delle protesi e degli ausili, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale in questione, al termine della sperimentazione, devono trasmettere una relazione alla Regione o Provincia autonoma recante l'elenco dei dispositivi erogati e una sintesi degli esiti. Questa previsione colloca il monitoraggio degli esiti a livello regionale, in quanto i medesimi saranno valutati solo a conclusione del previsto percorso di erogazione clinico assistenziale dei dispositivi in parola. Al riguardo si rammenta che l'articolo 104 dello stesso decreto del 2020, non essendo corredato da relazione tecnico-finanziaria, ha fin dalla fase istruttoria determinato problemi applicativi, esaminati anche in collaborazione con il MEF. Pertanto, è stato necessario richiedere un parere al Consiglio superiore di sanità, effettuare diverse interlocuzioni con il coordinamento tecnico dell'area assistenza territoriale della Commissione salute, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta in seno alla Conferenza Stato-Regioni. La disciplina specifica che regolamenta l'erogazione dei dispositivi sportivi per disabili va rinvenuta nel regolamento per l'erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all'avviamento alla pratica sportiva dei disabili di cui alla legge 27 dicembre 2017 e successivo decreto Le strutture già operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuabili sia nella banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili sportivi con le indicazioni dei relativi costi massimi ammessi rivolti a soddisfare le esigenze connesse all'avviamento dell'esercizio alla pratica sportiva, sia nella piattaforma *online* per consentire ai beneficiari di richiedere direttamente gli ausili sportivi da assegnare in comodato d'uso gratuito, avrebbero però sicuramente assicurato una procedura più snella di erogazione e di fruizione. L'attribuzione delle risorse sperimentali al Ministero della salute, più esigue di quelle assegnate al Dipartimento dello sport, ha invece determinato la necessità di risolvere una serie di complesse questioni attuative, al fine di delineare un *iter* di erogazione del tutto innovativo e inconsueto per le strutture di assistenza protesica regionali. Ne deriva che, coerentemente con la previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale in parola, le aziende relazioneranno alle Regioni sugli esiti della sperimentazione. Senatrice, come vede, non stiamo trascurando il *dossier*, che da Ministro e da medico considero parte non differibile della nostra missione. Le categorie fragili sono la nostra priorità, perché deboli e soprattutto perché, tutelando loro, potremo davvero dire di aver rispettato in pieno il mandato costituzionale.

il massimo del rispetto, non metto in dubbio la sua attenzione e la sua sensibilità, però le devo portare una Polaroid, una fotografia dello stato dell'arte. Lo so che il Ministero ha fatto quello che doveva, ma non ha raccolto poi sostanzialmente i *feedback* che comunque erano previsti nel decreto. Per mia personale esperienza e su mia personale sollecitazione a diverse Regioni, su venti Regioni ho avuto conferma e contezza che solo tre hanno di fatto emanato le delibere. Molte ASL territoriali non sono neanche a conoscenza del fondo. Ci sono tantissime persone con disabilità che, avendo io ovviamente negli anni pubblicizzato questa grande conquista - perché di fatto è stata tale -

se poi di fatto a cascata anche gli altri attori competenti non si adoperano per garantire e tutelare questo diritto a tutti, di fatto rimane marcata una discrepanza esagerata, che non si può più tollerare. Stiamo dicendo a tante persone con disabilità che lo sport è un lusso, quando dovrebbe essere un diritto, fermo restando che, al di là della scelta libera di praticarlo o meno a livello agonistico, è risaputo che la pratica sportiva, anche solo amatoriale, migliora lo stato di salute. Ministro, concludo velocemente e semplicemente chiedendole un'accortezza maggiore per un reale e concreto aggiornamento del nomenclatore. Dobbiamo smettere di guardare queste come voci di spesa: dobbiamo guardarle come investimenti a lungo termine, perché migliore è lo stato di salute anche di una persona con disabilità oggi, minore si presuppone sarà

finestra") *(M5S)*. Signor Ministro, il 14 febbraio 2024 il Ministero della salute ha emanato una circolare nella quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue, nella quale ha disposto alle unità di frontiera di intensificare i controlli sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia. Con il termine Dengue si intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere infettate dal virus Dengue, di cui esistono quattro diversi sierotipi. Più specificatamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo. La Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata anche Dengue emorragica, che può essere mortale. Tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo, ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta da due a sette giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara. Pertanto, anche gli emoderivati dovrebbero essere attenzionati.

Ciò premesso, chiedo di sapere da lei, signor Ministro, se sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti e scali merci) siano state già attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi previste nel PNA 2020-2025; se abbia già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

Con questa nota, nello specifico, sono state date disposizioni al fine di attuare, immediatamente e con prontezza, tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, con con riferimento specifico alla Dengue e alla prevenzione dell'introduzione della zanzara Aedes aegypty, principale vettore della malattia, attualmente non ancora presente in Italia. Ciò si è reso necessario per poter fornire pronta risposta all'aumento dei casi globali di Dengue soprattutto in Centro e Sud America e all'approssimarsi della stagione delle piogge nella fascia tropicale, e per garantire una maggiore sensibilizzazione nei riguardi dell'adesione alle necessarie misure di prevenzione. Desidero sottolineare che l'Italia si contraddistingue come il primo Paese europeo ad aver posto in essere immediatamente le misure di prevenzione della Dengue, attraverso l'azione del Ministero della salute e dei dipendenti degli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera collocati nei principali porti ed aeroporti italiani. Inoltre, l'Italia è tra i Paesi europei che hanno previsto, fin dall'epidemia della patologia zika in America meridionale e centrale, misure specifiche di disinfettazione degli aeromobili ai punti di ingresso e misure di igiene ambientale nei porti ed aeroporti. Per quanto concerne la dotazione del vaccino contro la Dengue, destinato all'utilizzo nell'ambito della medicina dei viaggi, preciso che in Italia è dispensato il vaccino denominato Qdenga. Allo stato attuale, il suo acquisto rientra nelle competenze dei servizi sanitari regionali. In merito alla segnalazione di casi sospetti, in applicazione del PNA 2025, la sorveglianza degli eventuali casi importati di malattia da virus Dengue nel territorio nazionale si estende per tutto l'anno, con la raccomandazione alle Regioni di potenziare il sistema di sorveglianza nel periodo di maggior attività vettoriale in termini di tempestività e sensibilità, per permettere l'identificazione rapida dei casi sospetti, per avere un'immediata e necessaria azione di controllo e per ridurre ogni rischio di trasmissione autoctona. Queste attività sono state effettuate anche nel corso della stagione vettoriale 2023. Sono stati registrati 362 casi di Dengue, 82 dei quali autoctoni. Questi dati sono in via di consolidamento. territorio nazionale sono stati identificati, al 21 febbraio 2024, 48 casi confermati di Dengue, tutti importati. Alla luce della panoramica illustrata, non posso che ribadire che la situazione in Italia oggi non risulta allarmante.

una settimana non mi sembra proprio che sia stata veramente data una risposta urgente. Detto ciò, effettivamente i casi - come lei ha affermato - sono molto di più di quegli 82 che ho citato, perché quelli erano solo gli autoctoni. Molto probabilmente nei casi non autoctoni si tratta di tratta di persone che sono andate a fare viaggi nei Paesi che hanno questo tipo di virosi, quindi sono passati proprio per gli USMAF e le unità territoriali, dove sostanzialmente viene presentato un documento per la vaccinazione. Vorrei rilevare che in questo documento con cui si dà il consenso per la vaccinazione la Dengue non viene proprio nominata. nominata. Vi invito veramente a rivedere il piano delle arbovirosi al fine di migliorare i protocolli per la raccolta delle informazioni sulla Dengue, nominando anche la Dengue in questo piano, soprattutto dando maggiori informazioni alla popolazione

questa volta parliamo di un trattato pandemico, mentre l'ultima volta parlavamo del regolamento pandemico. Cerchiamo quindi di fare un minimo di chiarezza per chi ci ascolta, perché sono cose molto diverse. Nello specifico, con trattato pandemico

Nella stessa data è prevista anche la possibilità di modifica del regolamento sanitario internazionale. Si tratta di due appuntamenti che, come parlamentare, ritengo ritengo molto importanti, perché stiamo parlando di due cose - una è un trattato internazionale e l'altra è un regolamento già in vigore - che diventerebbero sovraordinati al nostro ordinamento.

un'organizzazione in cui il peso dei privati sta diventando preponderante. Capite che i sospetti di conflitto d'interesse e quant'altro diventino molto problematici dal punto di vista di un legislatore. Vorrei sapere a che punto siamo con le negoziazioni e se è possibile intervenire a monte. Come abbiamo visto con il caso del MES - sono sempre tre lettere, ma alla fine l'arrivo è sempre quello - non vorremmo dover intervenire poi in sede di ratifica per dire di no in quella fase. Si può fermare prima? È una deriva che probabilmente porta a cose che sono auspicabili per l'OMS - per carità, le vogliamo tutti bene ma non necessariamente per gli Stati, per cui non vorremmo veramente essere costretti a dover fermare una valanga, quando si potrebbe fermare la palla di neve. Vorremmo quindi sapere a che punto sono le negoziazioni e se è possibile iniziare a far valere il nostro potenziale dissenso a monte, invece che a valle.

Al riguardo segnalo che nel dicembre 2021, in occasione della seconda sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità, i 194 Stati membri dell'OMS hanno determinato all'unanimità di stabilire un organismo di negoziazione intergovernativo finalizzato alla redazione e alla negoziazione di una convenzione, un accordo o altro strumento internazionale sulla prevenzione e preparazione in risposta alle pandemie. Parallelamente, è stato avviato un processo negoziale per la revisione del regolamento sanitario internazionale. L'avvio di quest'attività negoziale è stato oggetto della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 marzo 2022. La finalità di questi strumenti è quella di supportare gli sforzi internazionali volti a rafforzare i sistemi sanitari alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia, proprio partendo dalle criticità evidenziate nella gestione del Covid-19. Anche in più contesti internazionali multilaterali (il G7 e il G20), nonché europei, inclusi i *summit* più recenti, da ultimo in particolare il vertice G7 svoltosi a Hiroshima il 20 maggio 2023, è stato ribadito il supporto dei *leader* alla prosecuzione delle attività negoziali e al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero quello di avere strumenti rapidi, efficaci e più equi per rafforzare le capacità nazionali, regionali e mondiali, per consentirci di rispondere meglio nel caso in cui si verificasse un'altra emergenza sanitaria. Alla luce di quanto illustrato, evidenzio che l'Italia partecipa ai processi di negoziazione anche nell'ambito del coordinamento europeo, attraverso la rappresentanza permanente a Ginevra, con la collaborazione tecnica del Ministero della salute, assicurando la difesa e la tutela degli interessi nazionali, primi fra tutti i principi di equità, uguaglianza e universalità, che sono alla base dei nostri fondamenti costituzionali della tutela della salute. Infine, senatore Borghi, assicuro che il tema è presidiato e che le azioni, anche data la nostra Presidenza del G7, saranno in continuità con quanto già iniziato da questo Governo, della cui maggioranza anche lei è parte. Siamo in piena continuità con quanto il presidente del Consiglio Meloni ha già affermato in Giappone e in tutte le sedi non mancheremo di portare avanti gli interessi dell'Italia e degli italiani.

ma ricordiamoli, perché almeno devono essere chiari. Questo è un Governo che deve recuperare sovranità e non deve cederla. Un Governo che firma o si aggrega a trattati internazionali, che spesso e volentieri ci vedono parte minoritaria, non segue sicuramente i nostri interessi. Un Governo che si adegua a un regolamento che può essere infiltrato o colorato da interessi privati non fa i nostri interessi.

abbiamo inteso richiamare l'attenzione sua e del Governo su un tema di cui davvero siamo enormemente preoccupati: è un dramma che si chiama disuguaglianza, disparità nell'accesso al Servizio sanitario nazionale

territoriali evidenti già a partire dalla nascita, nonostante il Servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini. Eppure, queste disuguaglianze territoriali sono tanto accentuate che gli ultimi dati Istat disponibili ci parlano di tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita molto diverso: 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, il doppio in Sicilia e più che il doppio, purtroppo, in Calabria. Questi divari sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale: inutile richiamare la solita percentuale del PIL che ci vede molto al di sotto della Germania e della Francia, a fronte di un contributo privato comparativamente elevato e in Italia assai più elevato

e il privilegio di privati accreditati, a conferma di una volontà del Governo che sembra evidente, tesa a destrutturare il sistema sanitario pubblico. Colpiscono i dati sui livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle Regioni del Sud:

e Save the Children in questo rapporto ci dicono che con l'autonomia tutto potrebbe enormemente peggiorare, basta immaginare che le Regioni a statuto ordinario possono richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e quindi addirittura aprire una concorrenza tra loro al ribasso per il Mezzogiorno. È infatti il Mezzogiorno che soffre

e cinque delle otto Regioni del Mezzogiorno sono inadempienti, noi le domandiamo di spiegarci o di illustrare a noi e al Paese come si pensa davvero di rispondere alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali possano ulteriormente aumentare a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare una frattura difficilmente sanabile e profondamente ingiusta.

In via prioritaria e in estrema sintesi, osservo però che l'Italia non ha mai finanziato il Servizio sanitario nazionale con più del 7 per cento del PIL, con la sola eccezione del periodo del Covid. Non è possibile effettuare comparazioni tra i diversi Paesi utilizzando questo indicatore, che chiaramente dipende molto dalla ricchezza prodotta e non permette di apprezzare la dinamica del valore assoluto delle ingenti risorse messe a disposizione. Il sistema sanitario nazionale ha una matrice universalistica e, come chiarito dall'OMS in uno studio del 2009, ripreso recentemente dall'ufficio valutazione di impatto del Senato nel giugno scorso, i sistemi universalistici consumano il 3-4 per cento in meno di risorse per raggiungere pari livelli di salute. Questo impone attenzione, quando si fanno questi confronti internazionali. Il Ministero della salute è impegnato in via prioritaria a restituire ai cittadini un equo accesso alle cure per l'uniforme fruizione in tutto il territorio nazionale dei LEA da parte di tutti i cittadini della Nazione, cosa che negli anni passati non è sempre stata pienamente garantita. Quest'obiettivo strategico viene conseguito rinforzando da un punto di vista della dotazione finanziaria il nostro sistema, ma anche adeguando il modello di governo del rapporto fra Stato e Regioni. Per questo, come già anticipato, adotteremo un modello di programmazione sanitaria centrato sullo strumento del piano sanitario nazionale, che testimonia la volontà di passare da una *governance* pattizia (in questo caso, lo strumento è stato il patto per la salute) a una reale *governance* condivisa in cui Stato e Regioni si prendono responsabilità davvero condivise verso tutti i cittadini. Il piano sanitario nazionale non è un esercizio di stile, ma intende segnare un cambio di passo nelle relazioni tra livello centrale e regionale. Il cambiamento è reso possibile anche dalla capacità di utilizzare dati sempre più integrabili grazie all'investimento tecnologico dell'ecosistema dei dati sanitari. Questo permetterà di comprendere veramente il fabbisogno di salute, con un modello nazionale di classificazione e stratificazione dei bisogni, il relativo fabbisogno finanziario e di valutare le reali *performance* dei sistemi regionali, potendo così garantire il rispetto dei LEA. L'autonomia differenziata non mette in discussione l'unitarietà del diritto alla tutela della salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, come diritto e prerogativa di cittadinanza, così come declinato attraverso i LEA, ma rappresenta un potenziamento della facoltà delle Regioni di modulare la propria organizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei LEA, secondo le condizioni previste nell'articolo 116 della Costituzione. I LEA costituiscono in questa materia esplicazione della funzione di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Secondo quanto previsto nell'articolo 1 dello schema di disegno di legge in materia di autonomia differenziata, nella versione del 2 febbraio 2023, i LEA in sanità indicano una soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra Stato e autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. In quest'ambito, il Ministero della salute è fortemente impegnato nell'implementazione e nell'aggiornamento del contenuto delle prestazioni comprese nei LEA e nel rafforzamento dei relativi strumenti di *governance*. Ho pieno rispetto delle valutazioni Svimez, che da molti anni fotografano un'innegabile situazione di difficoltà delle Regioni del Sud, e vi posso garantire che non mancano gli sforzi per assicurare una piena attuazione dei LEA, indipendentemente dalla riforma sull'autonomia differenziata. Mi chiedo però se coloro che muovono le accuse di privatizzazione o di misure inconsistenti non siano gli stessi che invece di lavorare per l'abbattimento dei tetti di spesa per assumere personale hanno preferito negli anni precedenti che proliferassero le cooperative dei medici a gettone. Rivendico a questo Governo lo *stop* ai medici del gettone e il blocco dei tagli di questo Governo. Lo stanziamento di risorse per gli aumenti dei rinnovi contrattuali è un altro punto. Potevamo fare di più? Ovviamente sì, stiamo lavorando per farlo. Lasciate però tali ovvietà ad alcuni opinionisti, perché la visione su cui avete dubbi si realizza con la riorganizzazione delle strutture, con l'abolizione dei tetti di spesa, con lo scudo penale, con gli aumenti salariali e con gli incentivi per gli specializzandi, solo come alcuni esempi.

il nostro Servizio sanitario nazionale è ormai segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali e con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la frattura strutturale Nord-Sud. A questo, non rispondete e a chi ha dubbi sulle vostre responsabilità, dopo un anno e mezzo di Governo, suggerisco di toglierseli osservando cos'accade ad esempio in Abruzzo, dove governate da cinque anni. Lei stesso ha detto che ci dev'essere corresponsabilità tra Governo nazionale e regionale; mentre parliamo, proprio adesso, centinaia di persone esasperate hanno occupato l'ASL dell'Aquila contro lo sfascio della sanità pubblica. La Regione ha perso moltissimi reparti di eccellenza e paga 108 milioni di mobilità passiva, cioè in migliaia sono costretti a farsi curare in altre Regioni alle quali gli abruzzesi pagano i servizi e il personale, mentre i propri servizi e il proprio personale languono. Nei nostri ospedali mancano i più banali, ma fondamentali presidi sanitari: gli elettrodi per elettrocardiogrammi, i deflussori per flebo e addirittura i guanti monouso. Ancora, i pronto soccorso sono in continua emergenza, gli operatori sanitari sono esausti, le liste d'attesa sono ormai infinite e costringono gli utenti a rivolgersi ai privati oppure ad abbandonare le cure: lo fanno il 7 per cento dei cittadini e delle cittadine, evidentemente ormai di serie B, C o Z. Il personale assolutamente insufficiente è sempre più spinto ad abbandonare la nostra Regione verso sanità ben più accoglienti. È anche una chiara conseguenza del blocco dei tetti di spesa che non avete voluto affrontare e superare. Lei li ha citati: ricorderà che era il 2009 (Governo Berlusconi, Giorgia Meloni ministro). Assolutamente carente è l'edilizia sanitaria, con continui annunci di nuove strutture, che comunque sarebbero inutili senza nuovo personale, ma questo il romano Marsilio lo sa, visto che oltre a tornare ogni sera a casa sua, a Roma, si è guardato bene dal farsi curare e far curare i suoi cari nella sanità che lui stesso amministra. *(Applausi)*. E sa anche che l'autonomia differenziata per l'Abruzzo significa almeno 400 milioni di euro di trasferimenti in meno, che saranno tolti ancora alla sanità. È giusto che lo sappiano tutti i cittadini e i cittadini nel Mezzogiorno: questo è quello che vi aspetta, soprattutto dopo la cura dei patrioti secessionisti. Poi magari ci diranno: l'operazione è riuscita, il paziente è morto; ma noi glielo lo impediremo.

che ogni giorno ci sono a via Patini, per entrare nell'ufficio immigrazione della questura di Roma per la richiesta di asilo. Sono file lunghe, anche di 200 persone, che sono costrette a dormire davanti alla questura e a quell'ufficio, perché ogni giorno, secondo quanto ci risulta, la questura accetta solo dieci domande per quattro giorni alla settimana. Il diritto all'asilo è riconosciuto dall'articolo 10 della nostra Costituzione. È davvero indegno ed è dal 21 novembre che aspetto una risposta dal ministro Piantedosi su questa situazione, che non è solo di Roma.

La seduta è tolta